l'intendimento di rinviare il voto sul consiglio di amministrazione della Rai, anche alla luce del fatto - poi sicuramente ci sono altre considerazioni - che la Camera stessa

sono assolutamente contrario al rinvio del voto sul consiglio per due questioni. La prima riguarda la necessità di dotare l'azienda di una *governance* al più presto e di non lasciare in sospeso

l'altra questione che mi dà veramente fastidio è che tra i partiti che hanno richiesto il rinvio del CdA Rai c'è il MoVimento 5 Stelle. La ragione per cui non vogliono votare il nuovo consiglio di amministrazione è che non sono pronti in quanto il partito non è organizzato per dare un'indicazione: non hanno ancora chiaro se deve dare il nome Grillo o Conte.

Mi permetta, Presidente, di aggiungere una nota

oggi come non mai, in questo delicatissimo momento, che rischia di vederla schiantare per varie ragioni - anche di risorse che il Parlamento dovrebbe aumentare e riconoscere in quanto giuste. Non si

la Rai, così complessa e difficile da gestire, quando le forze politiche avrebbero potuto fare asse comune e proporre un nome interno (giravano vari nomi, uno dei quali era Del Brocco, una figura trasversale) o comunque il nome di una persona che conosca internamente i sistemi e i meccanismi di gestione della Rai.

intervengo solo per confermare che, pur apprezzando l'intervento del collega Faraone e i temi emersi, che ovviamente meriterebbe un dibattito molto più ampio,

siamo chiamati a convertire in legge il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che reca misure temporanee e provvisorie in attesa dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, relativa al riordino, alla semplificazione e al potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico universale. È una riforma epocale, quella di cui alla legge delega, di fondamentale importanza per tutte le famiglie di questo Paese, tanto importante che con il decreto-legge in conversione si è inteso anticiparne temporaneamente gli effetti, estendendoli anche in favore di nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Tale misura interviene temporaneamente - voglio ribadirlo, così come è stato ribadito dalla Commissione con l'approvazione di specifici emendamenti emendamenti - per dare un segnale di serietà e di vicinanza alle famiglie italiane in questa fase storica così complessa, ma senza voler in alcun modo allontanare la piena attuazione della delega da parte del Governo. una misura provvisoria, che al tempo stesso dà un segnale chiaro: sul sostegno economico alle famiglie l'Italia fa sul serio, promuovendo in modo attivo e concreto la genitorialità

di persone, famiglie, minori. Si tratta di un esempio di buona politica, di legislazione accurata e competente. Anche questo mi pare un dato importante, soprattutto se riportato al contesto della misura in esame e alla sua importanza. La misura temporanea e transitoria recata dal decreto-legge, erogabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, dunque per un periodo di sei mesi, consiste in un assegno mensile subordinato ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, il cui importo è determinato facendo riferimento al livello di ISEE e al numero dei figli minorenni. Come detto, l'assegno temporaneo in esame è disposto in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Ricordo che quest'ultimo è riconosciuto in presenza di determinate condizioni relative al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di figli minorenni, a condizioni di inabilità e con importi variabili, in favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla cosiddetta gestione separata INPS, dei titolari di trattamenti pensionistici o di altre prestazioni economiche previdenziali derivanti dalle suddette attività lavorative. L'assegno temporaneo, di cui agli articoli da 1 a 4, è riconosciuto qualora il richiedente possegga tutti i requisiti di cui all'articolo 1 e limitatamente al periodo in cui essi sussistano. La domanda per l'assegno temporaneo in esame è presentata in modalità telematica all'INPS, ovvero agli istituti di patronato e di assistenza sociale, secondo le modalità indicate dall'INPS, entro il 30 giugno 2021. L'assegno, nell'ambito del periodo temporale massimo di applicazione (costituito, come detto, dal secondo semestre 2021), decorre dal mese di presentazione della domanda con il diritto, tuttavia, alle mensilità arretrate per le domande presentate entro il 30 settembre 2021. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente, ovvero mediante bonifico domiciliato. Nel caso di affidamento condiviso del minore in relazione al quale sia corrisposto l'assegno, la metà dell'importo può essere accreditata sul conto corrente bancario o postale dell'altro genitore. L'assegno in esame non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è compatibile con altre eventuali prestazioni in favore dei figli a carico erogate dalle Regioni o Province autonome e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla citata legge n. 46, con le misure, ad eccezione del summenzionato istituto dell'assegno per il nucleo familiare, familiare, indicate nell'articolo 3, comma 1, di questa legge. Per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, il beneficio temporaneo in oggetto è corrisposto nell'ambito del summenzionato limite massimo complessivo di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, di ufficio dall'INPS ad integrazione del reddito di cittadinanza e con le medesime modalità di erogazione di quest'ultimo. In ogni caso, l'assegno temporaneo in esame è escluso dalle nozioni di reddito familiare assunte a base del calcolo dell'imposta sul reddito di cittadinanza. L'articolo 5 dispone in via transitoria, per il periodo che decorre dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. L'incremento concerne solo i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e per i nuclei familiari con almeno tre figli a 55 euro per ciascun figlio. L'articolo 6 dispone per il 2021 un incremento nella misura di 30 milioni di euro del finanziamento statale per la convenzione tra INPS e i centri di assistenza fiscale, in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche. L'articolo 7 reca alcune norme in materia di finanziamento, nonché di relativo monitoraggio finanziario, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19. L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento. Colleghe e colleghi, riferisco oggi a questa Assemblea gli esiti del lavoro faticoso svolto dalla Commissione, nello svolgimento del quale siamo stati guidati dalla consapevolezza di alcuni punti fondamentali che qui voglio ribadire: innanzitutto la temporaneità della misura e l'assoluta necessità di procedere parallelamente alla sua erogazione, alla rapida attuazione della delega di cui alla legge n. in secondo luogo, la forte attenzione al sostegno alla genitorialità; in terzo luogo, abbiamo percepito con chiarezza, in sede di approfondimento in Commissione, alcune criticità relative soprattutto alla forte progressività a cui sono ispirati i criteri di individuazione della soglia ISEE, con la conseguente diminuzione proporzionale dell'importo dell'assegno al miglioramento della situazione economica del nucleo familiare. Siamo consapevoli che ciò può determinare il rischio di disincentivare il lavoro del secondo percettore di reddito del nucleo familiare, coincidente, nella maggior parte dei casi, con le donne. Proprio per questo, pur non intervenendo direttamente in Commissione, è stato depositato un ordine del giorno che impegna il Governo a farsi carico, in sede di attuazione della delega, di tale questione, soprattutto al fine di dare piena attuazione alla finalità espressa dall'articolo 1 della legge n. 46 di promuovere l'occupazione ed in particolare quella femminile. Stiamo ragionando, colleghe e colleghi, di una misura temporanea e allo stesso tempo, come detto, stiamo dando un segnale di grande serietà e di vigilanza a tutte le famiglie italiane. Sono convinto che il lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge su cui riferisco all'Assemblea abbia consentito di approfondire snodi essenziali e potenziali criticità della stessa disciplina che dovrà essere adottata in attuazione della delega. Anche questo consegniamo oggi all'Assemblea. Su tutto, però, colleghe e colleghi, siamo stati guidati dalla certezza di svolgere un lavoro importante per dare alle famiglie italiane e alla genitorialità un sostegno immediato, concreto, fondamentale in una fase come questa e di ciò possiamo dirci orgogliose ed orgogliosi.

la conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Ci ritroviamo quindi a dover operare una scelta, più o meno condivisa, su un provvedimento che pensavamo di

Lo dico perché è importante che le cose vengano chiamate con il loro nome. Ciò si evince anche all'interno del testo, nelle indicazioni dei requisiti.

provvedimento di sostegno al reddito. La particolarità di questo, però, sta nel fatto che, mentre nel disegno di legge delega, che chiaramente è diventato legge, assistiamo a un accorpamento di fondi e quindi alla mancata possibilità per alcuni nuclei di usufruire di sgravi fiscali, in questo caso tale accorpamento non viene fatto.

ma in maniera tale che vi sia una prospettiva di investimento, cioè che le quote vengano investite sul territorio italiano, creando un circolo virtuoso sul piano macroeconomico. Anche questo non è stato assolutamente tenuto in considerazione. È stato accolto l'ennesimo ordine

dettagliato meglio un termine di novanta giorni, qualora il Governo lo assuma per intero, entro cui vagliare questa modifica dell'ISEE.

scenderà - se non si inverte la tendenza - a circa 30,5 milioni di persone. Le Camere, da tempo, sollecitano l'attenzione verso il progressivo dimezzamento in atto della popolazione in Italia, a causa della crescita zero, con conseguente invecchiamento più veloce da noi che nel resto d'Europa. Forza Italia è da sempre favorevole alle iniziative politiche, sociali ed economiche che sono indirizzate al sostegno delle famiglie, ad una riforma del sistema fiscale che sia di sostegno alle stesse e conseguentemente alla natalità, che va difesa e incentivata con interventi specifici di lungo periodo. L'assegno unico e universale è una di queste misure di sostegno che potrebbero aiutare la natalità italiana, se naturalmente la sua attuazione avvenisse in un contesto di crescita economica, di occupazione, di riduzione del tempo di precariato, di riorganizzazione della spesa pubblica indirizzata ai minori e di diminuzione del prelievo fiscale. Il decreto-legge in esame rappresenta la misura ponte dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti per ogni figlio minore di diciotto anni, inclusi i figli minori adottati o in affido. Riguarda le famiglie in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 50.000 euro annui, fino all'entrata a regime dell'assegno universale e unico per ogni figlio, che avverrà a decorrere dal gennaio 2022. Gli oneri di spesa previsti per l'anno 2021, per gli articoli 2, 5 e 6, sono pari a 3 milioni di euro. Con il provvedimento in esame, l'assegno temporaneo viene corrisposto alle famiglie con figli minori che, in base alla legislazione vigente, non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare. L'assegno viene erogato in funzione del numero dei figli, per cui gli importi dell'assegno decrescono all'aumentare dell'ISEE e sono più elevati per le famiglie con tre o più figli. L'assegno da erogarsi si azzera raggiunta la soglia dei 50.000 di ISEE. L'assegno temporaneo è pagato mensilmente dall'INPS sulla base della domanda presentata. Le audizioni dell'11a Commissione hanno fatto emergere alcune criticità dell'impianto normativo del decreto-legge, che ritengo possano indebolire il principio universalistico a cui il decreto-legge vorrebbe tendere: innanzitutto, la soglia dei 50.000 euro dell'ISEE, rispetto a quegli Stati, anche europei, con forti politiche di sostegno alla natalità, dove l'aver figli è considerato una scelta personale, nell'interesse della Nazione, misure simili non vengono proporzionate in relazione al reddito familiare, in quanto l'indicatore ISEE penalizza i redditi familiari rispetto a quelli individuali e l'utilizzo dell'ISEE rischia di determinare effetti distorsivi e sperequativi, in particolare per determinate categorie di cittadini. È stato fatto osservare che per l'assegno unico universale il ricorso alla sola componente reddituale dell'ISEE per la definizione del beneficio in luogo dell'intero indicatore sarebbe di gran lunga preferibile. La progressività molto rapida, che dimezza l'importo dell'assegno, disincentiva le famiglie con reddito contenuto ad aumentarlo. l'accentuazione del beneficio nei confronti delle famiglie con almeno tre figli: com'è stato fatto rilevare dal mondo delle imprese, garantire un assegno mensile cumulabile con la misura del reddito di cittadinanza potrebbe comportare il verificarsi di paradossali situazioni, nell'ambito delle quali le imprese si trovino in ancor più difficoltà nella ricerca di forza lavoro, configurandosi la concreta possibilità che lo stipendio medio garantito dell'impresa sia inferiore rispetto al sussidio garantito dallo Stato e che dunque questa misura agisca come possibile disincentivo all'occupazione. Per migliorare l'efficacia del provvedimento, Forza Italia ha deciso di presentare alcuni emendamenti riconducibili all'ISEE, che non sono stati resi ammissibili ai sensi dell'art. 81 della Costituzione. Non per fatto personale, credo che sia necessaria una seria riflessione sull'utilizzo dell'articolo 81, nel senso che talvolta non appare assolutamente chiara la criticità finanziaria che un emendamento determina. Gli emendamenti che abbiamo proposto intervengono, in particolare, sulle soglie ISEE, al fine di computare per il calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente del nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento. Inoltre, riteniamo che il possesso di una sola abitazione dove la persona o la famiglia vive non debba essere considerato elemento che possa inficiare il diritto ad avere certe prestazioni sociali in quanto il bene determina una crescita del proprio indicatore della situazione economica. Malgrado la bocciatura delle nostre proposte emendative, Forza Italia, che è sempre attenta nei confronti di proposte legislative che riguardano le politiche per la famiglia e per i figli, ritiene comunque di esprimersi a favore del provvedimento in esame.

rappresentante del Governo, colleghi, finalmente ha trovato attuazione l'articolo 3 della nostra Costituzione, con la parificazione delle diverse categorie di cittadini italiani. Infatti, con questo provvedimento si mette fine alla discriminazione fra lavoratori dipendenti e autonomi, dato che i secondi ora potranno percepire l'assegno per i figli a carico. il progressivo abbassamento del tasso di natalità degli italiani, si rendono necessarie nuove leggi per incoraggiare la fecondità dei nostri giovani. Ufficialmente anche la legge oggi in discussione e valida fino a fine anno dovrebbe farlo, ma penso che l'esiguità degli assegni previsti con questo metodo di calcolo penalizzi, invece, la natalità degli italiani. Essa crea aspettative piuttosto onerose per i futuri bilanci, se anche il provvedimento che andrà a regime dal prossimo anno seguirà le medesime orme. Infatti, se una coppia di giovani, entrambi lavoratori, desiderasse avere figli, è molto facile che l'ISEE risultante sia vicina a 40.000-50.000 euro e l'assegno pensato per incoraggiare la loro genitorialità ammonterebbe solo a 30-40 euro al mese, davvero troppo poco per incentivarli in questo senso, anche perché un asilo nido costa mediamente sui 6.000-7.000 euro all'anno. Invece, una coppia con ISEE basso o priva di reddito, avendo cinque figli a carico, arriva a percepire 1.089 euro mensili, da sommare poi anche il reddito di cittadinanza, quindi potrebbe verificarsi la concreta possibilità che il sussidio garantito dallo Stato sia superiore allo stipendio medio garantito da un'impresa qualsiasi. Questa legge, perciò, potrebbe concretamente disincentivare la ricerca di un lavoro. Se davvero l'Italia volesse incoraggiare la natalità di suoi concittadini, potrebbe essere molto più utile che il costo della maternità fosse fosse interamente a carico dello Stato, senza oneri per i datori di lavoro, compreso anche lo sgravio contributivo per il personale in sostituzione delle lavoratrici in maternità. Quanto sopra, se aggiuntivo a un buon sistema di *welfare*, all'accompagnamento e all'inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro, offrendo loro stabilità lavorativa ed economica, costituirebbe un vero e proprio volano per una robusta natalità nel nostro Paese. Per restare al provvedimento oggi in esame, mi pare che il grosso peso dell'ISEE nella distribuzione dell'assegno crei forti disparità di trattamento fra bambino e bambino. Questo non accade in altri Paesi europei che hanno adottato idonee politiche per incentivare la natalità, come in altri Paesi non è riconosciuto l'assegno per i figli minori agli stranieri extraeuropei privi dello *status* di rifugiato politico

legge, pertanto, più che incentivare la natalità degli italiani, mi sembra l'ennesimo provvedimento assistenzialista contro la povertà: penso che siamo proprio un Paese buono e magnanimo. Peccato che la spesa di tutto ciò sia a *deficit* e a carico delle future generazioni di italiani e che, proprio con questo provvedimento, corriamo il rischio che non ne nascano a sufficienza. *(Applausi)*. Signor Presidente, l'Italia attraversa un periodo ormai molto lungo di denatalità:

nascevano più bambini in Italia quando gli italiani erano meno di 40 milioni, appena arrivati all'Unità del nostro Paese, di quanti ne nascano oggi. Ne nasce poco più di un terzo del periodo in cui sono nato io, e questo nonostante il fatto che

resteranno a quel livello, con tutti i riflessi che questo avrà sulla nostra forza lavoro, sugli aspetti previdenziali e anche sull'andamento generale della società.

però sono uomini - si ridurranno quando questo grosso calo di natalità arriverà all'età fertile.

sempre più breve durata media dei matrimoni o delle relazioni di coppia (anche questo, a seconda della Costituzione, che probabilmente si vorrà aggiornare, è

con una certa rilassatezza: naturalmente, con attenzione al bilancio familiare, può anche pagarsi qualche lusso, qualche vacanza e qualche uscita al ristorante. Se questa stessa coppia ha uno o due, per non parlare di tre figli (che tra l'altro è il numero che può garantire l'equilibrio della popolazione: considerate tutte le coppie o persone che non hanno figli, è davvero il numero indispensabile), indispensabile), siamo sulla soglia della povertà: le persone devono misurare il centesimo, perché lo Stato oggi dà alle coppie con figli - sempre che dia qualcosa in termini di detrazioni fiscali, perché al di sopra di un certo livello, molto basso, non dà assolutamente nulla assolutamente nulla - molto meno di quanto incassa in più per tutto ciò che si deve comprare quando si hanno bambini, dalla culla, al lettino, all'auto più grande (perché una coppia può avere un'auto piccola, mentre una che abbia due figli ha bisogno di un'auto e di una casa più grandi). È un cattivo affare avere figli, in un'epoca in cui già c'è una difficoltà economica generalizzata. Dunque ben venga l'assegno unico universale. Bellissimi il nome

euro al mese. Ciò evidentemente non induce nessuna coppia ad avere figli. È sempre meglio di niente, ma il problema non è che oggi non ci sia niente: l'anno prossimo queste misure saranno anche sostitutive di altre, pure insufficienti, che oggi ci sono.

la Lega ritiene che l'oggetto di questo provvedimento e di questo dibattito sia di fondamentale importanza per il futuro del nostro Paese e della nostra società. Parliamo di assegno unico universale per i figli minori a carico, quindi di uno strumento che deve tutelare la famiglia, soprattutto se decide di avere figli. In una società come la nostra, in cui la denatalità è un problema sempre maggiore, con dati che non vanno migliorando negli anni, anzi peggiorando, è evidente che un intervento della politica, del Parlamento e del Governo si rende assolutamente necessario ed è indispensabile.

dicembre di quest'anno, con l'introduzione di un assegno temporaneo per i figli minori. Questo a fronte della misura approvata nei mesi scorsi, che invece vuole istituire con delega al Governo un assegno unico universale, che andrà a realizzarsi a partire dal prossimo anno e per quelli a venire. Si tratta quindi di un provvedimento temporaneo e sperimentale che dev'essere solo propedeutico a una riforma più complessiva.

puntare la nostra attenzione. Il provvedimento approvato di delega al Governo stabiliva di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli. Il Gruppo Lega chiede effettiva garanzia che, quando si parla di riordinare e semplificare, ci sia un effettivo potenziamento delle risorse messe a disposizione e della loro efficacia.

una certa abitudine a diffidare del termine semplificazione. Spesso in quest'Aula si portano avanti provvedimenti che parlano di semplificazione e che alla fine non rappresentano un miglioramento, ma in alcuni casi, per alcune categorie e, in questo caso, per alcune famiglie, potrebbero rappresentare un peggioramento. Vigileremo su questi aspetti e ovviamente sui decreti attuativi del Governo affinché ciò non accada.

Per chi ha un reddito ISEE superiore a 50.000 euro non c'è nulla. Anche nella fascia tra i 15.000 e i 50.000 euro parliamo di 30 euro mensili

realtà dei fatti. Ci sono pertanto risorse che dal nostro punto di vista sono inadeguate. Ci auguriamo quindi che le risorse che verranno stanziate successivamente, a partire dal prossimo anno, siano potenziate e rappresentino un effettivo aiuto alle famiglie e non solo

che ci sia una rivisitazione dei criteri ISEE che non sempre rappresentano l'effettivo benessere delle famiglie e che ci siano risorse adeguate, che non rappresentino un palliativo a un problema ben più ampio. Questa è la sfida che ci aspetta come Parlamento, ma che ovviamente riguarda soprattutto il Governo. Da parte nostra, non potremo far altro che vigilare, il principio è corretto, ma la risposta dev'essere assolutamente adeguata e conforme alle aspettative della nostra cittadinanza. Le famiglie si trovano in una grave crisi e tutti dobbiamo esserne consapevoli. Il tema meriterebbe molta più attenzione e approfondimenti di quelli di attualità che, invece, altri partiti vogliono mettere al primo posto nell'agenda politica,

e di coloro che svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società. La Lega su questi temi c'è e vigilerà perché le risposte del Governo siano adeguate. *(Applausi)*.

non è soltanto pensando alle nostre drammatiche politiche demografiche per cui siamo un Paese a crescita zero

è anche pensando al forte collante che nella vita di famiglia costituisce la possibilità di mantenere tra i coniugi e le persone che compongono il nucleo familiare quel minimo livello di serenità e di positività che fa sì che la benedetta fatica del lavoro quotidiano, quando c'è, possa aprirsi anche a uno sguardo di speranza per il futuro per poter offrire ai figli qualcosa di più che non sia lo strettamente necessario.

Proprio perché crediamo nel valore di una misura positiva che vada incontro alle necessità delle famiglie e a quella specifica dei figli, riteniamo che questa corra il rischio di essere una misura *spot*.

(penso a coloro che ricevono un reddito di cittadinanza e che, con mio stupore, non devono nemmeno fare la domanda, perché viene loro accreditato in automatico, senza doversi prendere la briga

Probabilmente sono una cifra significativa. Ognuno di noi, se esce con un amico una sera per un *happy hour*, spende 37 euro; probabilmente, se due ragazzi escono, come ieri sera, per festeggiare

un incentivo alla natalità? In che modo un genitore può sentirsi incoraggiato ad avere un figlio? Conosciamo l'aneddoto che dice che tutti vorrebbero avere tre figli; poi si sposano e ne vorrebbero due, possibilmente un maschio e una femmina, sempre facendo riferimento a identità ben consolidate, e poi invece si accontentano di un unico figlio, perché non riescono a mantenerne di più.

dall'altra, la totale e assoluta inadeguatezza della misura rapportata ai bisogni. E sappiamo che, quando non sono esigibili,

Mentre la misura economica viene da una povertà che attualmente rende molto basso il reddito percepito e quello realmente ottenuto,

ma se queste non si trasformano in una fattualità concreta, dall'illusione scaturisce la delusione, e questo può essere molto pericoloso per le nostre famiglie.

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, signori e signore del Governo, il provvedimento che stiamo per approvare è frutto di un lavoro molto lungo, nato da una proposta di Italia Viva e già riconosciuto dal precedente Governo. La conversione di questo decreto-legge permette una vera e propria riforma rivoluzionaria che il Paese attende da anni e che arriva in un momento in cui è estremamente necessaria per sostenere le famiglie italiane e aiutarle a progettare la ripartenza dopo la drammatica crisi causata dalla pandemia. L'assegno unico è un grande pezzo del più grande e generale *family act* che il Governo ha approvato e che da qui a qualche tempo anche il Parlamento discuterà. Com'è noto, esso mette a disposizione risorse finanziarie dal settimo mese fino ai diciotto anni di età; si estende fino ai ventun anni quando ci sono attività importanti di formazione ed educazione e ha una specifica formulazione anche in termini di indicazioni finanziarie per i figli che hanno problemi di disabilità. È una misura che offre un contributo importante, che va da 168 euro a figlio fino a 217, se ne hanno più di due. Ad oggi, a sette giorni dal via, sono arrivate più di 150.000 domande. Si può richiedere l'accesso al beneficio fino al 30 settembre prossimo, prendendo gli assegni arretrati dal 1° luglio scorso. Questo grande numero di domande pervenute ci fa capire tutta la bontà della norma che abbiamo fortemente voluto. Al centro dell'azione del provvedimento, quindi, vi è finalmente la famiglia. Italia Viva e questo Governo hanno finalmente - e sottolineo l'avverbio, signor Ministro - messo la famiglia al centro non solo dell'azione dell'Esecutivo, ma anche dello sviluppo delle politiche demografiche del nostro Paese. Dal 1945 ad oggi, infatti, le nascite si sono dimezzate. L'Istat negli ultimi dati presenta cifre clamorose: poco più di 400.000 nati annui contro circa 700.000 deceduti. In questo saldo naturale così negativo, è evidente che, senza interventi urgenti per il nostro Paese, ci sono all'orizzonte solamente prospettive difficili di sviluppo e di crescita. Grazie all'assegno possiamo invertire il pauroso fenomeno del dimezzamento delle nascite e metterci in carreggiata con i Paesi più attrezzati in tema di politiche familiari, proponendoci finalmente come terra ospitale per i giovani, per le giovani coppie e per le famiglie che vogliono continuare a credere e a investire nel futuro. L'Italia è un Paese che ha costruito, nel corso degli anni, tantissime agevolazioni di tipo fiscale: sono circa 500 quelle che vengono censite, ma di queste pochissime sono state dedicate o sono dedicate alla famiglia. L'assegno è unico, perché riorganizza una giungla di misure, bonus e detrazioni stratificate nel tempo. Semplifica la vita delle famiglie e alle famiglie, permettendo loro di ricevere una misura di programmazione e di stabilità nel tempo. È un provvedimento attivante, come spesso diciamo, perché stimola la famiglia a proiettarsi nel futuro e a compiere scelte coraggiose. Le politiche familiari danno i frutti migliori quando hanno un carattere di stabilità, perché danno un'autonomia nella progettazione economica della vita. Grazie all'assegno unico, ogni mese una famiglia saprà di poter contare su un importo fisso fino ai ventun anni di età di ciascun figlio. Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione per il nostro Paese. Dovremmo poter consentire alle stesse famiglie di richiedere l'attivazione dell'assegno universale, oltre che all'INPS e ai CAF, anche tramite i patronati - l'ho detto già precedentemente - che sono al momento esclusi e che - mi permetto di dire - in questo momento particolare si sono spesso gratuitamente sostituiti al lavoro dell'INPS. È un investimento sullo sviluppo sociale, che non rende le famiglie dipendenti da un aiuto *spot* dello Stato, come altri inutili provvedimenti assistenziali. Italia Viva dimostra di essere ancora una volta un grande movimento riformista, che non propone misure *spot* e senza visione; è invece un luogo sano di presentazione di proposte concrete e realizzabili per il futuro del nostro Paese. Noi abbiamo a cuore l'Italia del domani, un'Italia che, grazie al contributo determinante del ministro Elena Bonetti, a cui va tutta la nostra gratitudine per il lavoro costantemente ed efficacemente svolto, e grazie al lavoro di questo Governo,

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, egregi colleghi, il tema che oggi stiamo dibattendo in quest'Aula è di fondamentale importanza, perché parla - e ciò accade proprio raramente - di futuro. Parla del futuro delle generazioni più giovani di noi, che avranno l'onore e l'onere di essere parte integrante della nostra società. Viviamo in una società oggi condizionata purtroppo da falsi miti; le giovanissime generazioni venerano personaggi televisivi, cantanti musicali o *star* dei *social* in base al numero di *follower* su Instagram o Facebook. I miti veri, colleghi, in una società come quella di oggi, sono invece quegli *under* 40 che hanno la capacità di compiere il gesto più rivoluzionario che si possa fare oggi: costruire una famiglia e dare ad essa Queste sono le persone a cui i giovanissimi di oggi dovrebbero ispirarsi; e noi, che facciamo politica in modo serio, abbiamo il compito di sostenerle. Tuttavia - e di certo la pandemia non ha aiutato - viviamo un periodo storico in cui per le giovani generazioni il lavoro è sempre più precario, la casa un lusso e la pensione un miraggio che mai si concretizzerà. Intervenire oggi, quindi, con uno strumento legislativo che possa aiutare le famiglie è un bene. È arrivato il momento di smentire quel detto popolare, vero purtroppo, in cui si dice che durante la guerra gli italiani stavano peggio di adesso eppure mettevano al mondo molti più bambini. Questo è dovuto al fatto che fortunatamente in una famiglia prevalgono spesso le motivazioni culturali per cui si fa un figlio rispetto a quelle materiali. Tuttavia è innegabile che oggi le condizioni sono molto cambiate: mettere al mondo un figlio richiede molte più risorse, poiché la società in cui viviamo oggi non ci non ci permette di crescere un bambino vestendolo di stracci e nutrendolo con una scodella di latte e pane. Per questo, colleghi, con lo sviluppo della società moderna gli Stati hanno incominciato a porsi il problema di aiutare le famiglie a mantenere i figli e l'Italia nei decenni scorsi non ha di certo brillato. È noto a tutti che il nostro Paese è uno di quelli con il tasso di fecondità più basso al contempo, è tra quelli che destinano meno risorse per famiglia e figli. Questa è una contraddizione, poiché ovviamente, se si vogliono aiutare le famiglie, bisogna investire Secondo i dati Eurostat mediamente riusciamo a destinare il 3,2 per cento della spesa pubblica italiana alle politiche familiari, contro il 3,6 per cento della media europea:

visto che negli ultimi anni i loro investimenti non arrivano al 2 per cento. Di contro (ma di certo non si vuole creare un conflitto tra giovani ed anziani), siamo ai primi posti quanto a uscite per la previdenza pensionistica, il che significa il 32,8 per cento della spesa pubblica contro il 26,4 per cento della Francia, cento della Germania, il 21,4 per cento della Svezia, il 16 per cento della Danimarca. Ben venga quindi, cari colleghi, l'assegno unico come strumento di aiuto nei confronti delle giovani generazioni, purché esso non sia considerato una forma di contrasto alla povertà, verso la quale si dovrebbe intervenire in altri modi, sicuramente migliori rispetto al reddito di cittadinanza, ma un intervento a beneficio dell'investimento sui figli, considerati un bene pubblico. Dando un rapido sguardo ad alcuni Paesi europei, scopriamo che in Francia spettano circa 130 euro al mese con il secondo figlio, in Germania circa 200 euro al mese per ogni figlio, nel Regno Unito 100 euro al primo figlio al primo figlio e 60 ai successivi, in Svezia 100 euro a figlio più *bonus,* in Olanda 100 euro a figlio. Dobbiamo poi anche preoccuparci delle storture che alcune miopi politiche sociali producono in Italia. Le poche risorse che il nostro Paese destina ai figli producono famiglie con redditi bassi, che si avvicinano alla povertà relativamente al numero dei figli. Possiamo quindi sostenere che l'Italia è un Paese che disincentiva la natalità, pertanto anche noi siamo dell'idea che sia doveroso intervenire su questo tema, ma ciò non impedisce in alcun modo di sottolineare cosa potrebbe essere migliorabile. Secondo il decreto-legge sarà l'INPS, infatti, a gestire l'implementazione dell'assegno unico temporaneo, al quale dovrà essere inoltrata la domanda per l'assegno ponte, di cui beneficeranno circa 1,8 milioni di famiglie. L'obiettivo condivisibile è quello di un sistema universalistico, di cui beneficeranno lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti, incapienti e molte altre categorie. Il rischio, come è emerso dalle audizioni fatte dalla 11a Commissione, è una non equilibrata distribuzione degli effetti di cui si dovrà tenere conto in fase di implementazione della riforma; una riforma che sembrerebbe voler mantenere in vigore alcuni istituti vigenti, creando non poca confusione alla famiglia che vorrà accedere a questi sostegni. Un altro aspetto che vorremmo considerare è legato a come diminuire la differenza di sostegno tra i lavoratori autonomi e quelli subordinati. L'esperienza di quest'ultimo periodo, legata alle difficoltà dovute alla pandemia per il Covid, ha fatto emergere con chiarezza l'inaccettabilità di politiche di sostegno al reddito spesso indirizzate in modo asimmetrico a lavoratori subordinati. Alcuni dati che ci sono stati forniti in Commissione evidenziano come i lavoratori autonomi hanno registrato la diminuzione più consistente dei redditi familiari dall'inizio della crisi: per cento ha infatti registrato un calo del reddito e nell'8,8 per cento dei casi la perdita è stata ad un livello superiore al 50 È un dato di fatto che nel campo del lavoro autonomo ci sono state differenze nei livelli di copertura forniti dalle misure di sostegno messe in campo dal Governo, nonché differenti modalità di accesso alle stesse, che hanno visto sistematicamente penalizzati i lavoratori autonomi: è questa una problematica cui è doveroso porre rimedio. Anche le risorse meritano una riflessione, perché anche a regime non consentiranno di ottenere l'obiettivo di un assegno medio mensile prossimo ai 250 euro per ogni figlio, fino a ventuno anni di età, come annunciato dal presidente Draghi ispirandosi ad altri Paesi dell'Unione europea. Anche se i valori sono qualitativamente apprezzabili per i benefici, riduce in modo significativo l'impatto della riforma e la sua pretesa di universalità. In quasi tutti i Paesi europei che hanno avanzate, importanti e convinte politiche di sostegno alla natalità, viene rilevato che queste stesse misure non vengono proporzionate in relazione al reddito familiare perché il rischio è che l'utilizzo dell'indicatore ISEE per delimitare il numero dei beneficiari dell'assegno unico produca di fatto l'effetto di penalizzare i redditi familiari rispetto a quelli individuali. In Francia, ad esempio, è stato introdotto il quoziente familiare che suddivide una parte del reddito tassabile e relativa aliquota di prelievo in rapporto ai carichi familiari, ottenendo esattamente l'effetto opposto all'ISEE. Infine, colleghi, esprimo un'ultima perplessità: i nuclei composti da cinque componenti, di cui tre figli minori che già percepiscano il reddito di cittadinanza e possiedano un ISEE che si attesta intorno ai 7.000 euro potranno arrivare complessivamente a ricevere 1.653 euro mensili, ben 19.800 euro all'anno, cifra destinata ad elevarsi ulteriormente qualora la famiglia risieda all'interno di una casa in affitto e abbia diritto al contributo di 200 euro previsto. Infine, ciò è sicuramente positivo in una logica assistenziale, ma potrebbe costituire un deterrente ad un comportamento attivo nella ricerca di una occupazione: guai ad incappare nella morsa dell'assistenzialismo che non abbia un fine e un progetto legato al futuro. Per noi di Fratelli d'Italia sarebbe un imperdonabile errore nei confronti di quelle tantissime famiglie che sognano una famiglia compatibile con un'appagata crescita professionale e sociale.

questo decreto cosiddetto ponte, di natura transitoria per l'assegno unico universale ci debba accompagnare positivamente verso la piena ed importantissima riforma che andrà a regime dal 1° gennaio 2022.

perché l'assegno unico e universale allinea l'Italia alle migliori esperienze europee. Credo che questa sia stata una scelta molto importante. un assegno unico e universale: unico perché va a sostituire, come abbiamo detto, tutte le attuali forme di sostegno alle famiglie *bonus* bebè, *bonus* mamme, *bonus* terzo figlio); universale perché sarà corrisposto ogni mese a tutti, senza distinzione tra lavoratrici e lavoratori dipendenti, autonomi, capienti e non capienti, con una maggiorazione per chi ha figli con disabilità. Era ed è una riforma attesa dal Paese, necessaria, positiva, che - lo voglio dire - il Partito Democratico ha promosso fin dalla scorsa legislatura, rispetto alla quale poi siamo tornati tutti ad essere convinti; una riforma che semplifica un sistema complesso e composito, chiude la stagione dei *bonus* a pioggia e introduce uno strumento strutturale, sicuro e continuo per venire incontro ai bisogni delle famiglie.

italiano, anche perché, da questo punto di vista, noi includiamo ogni tipologia di famiglia, anche le famiglie povere. Questo è il punto, perché mettiamo al centro i bambini, i figli e le figlie. a mio avviso, un elemento particolarmente importante, anche perché voglio sottolineare che la scelta dell'assegno unico e universale colma un vuoto e segna un profondo cambiamento del nostro *welfare* e della cultura in base alla quale si è costruito

risorse dedicate e distribuite in modo diverso da modelli precedenti e, tra l'altro, da questo punto di vista anche particolarmente efficaci. Quindi, questa riforma unisce, secondo noi, alla concretezza le risorse. Certo, bisogna mettere risorse adeguate per completare e compiere effettivamente questa riforma, che va verso il senso universale della rete di protezione sociale.

che si è svolta sul disegno di legge, il *family act*, in cui si inizia a discutere della condivisione del lavori di cura. Dico tutto questo perché, se l'assegno unico universale non lo collochiamo all'interno di una visione di sistema, di rilancio della centralità dell'occupazione femminile, rischiamo di

al secondo percettore di reddito, perché altrimenti si rischia una contraddizione sull'impianto e sulla finalità della riforma. Facciamo attenzione a questo aspetto. Prevalentemente,

che sarebbe dovuto entrare in vigore fin dallo scorso 1° luglio con ben altre prospettive. Quest'ultimo rappresenta infatti una misura proattiva che assorbe gli esistenti assegni familiari e le detrazioni, quindi è volto anche ad un sistema di semplificazione ed è rivolto ad una platea più vasta rispetto a quella che percepirà l'assegno ponte. Questa misura invece è un provvedimento a sé stante, transitorio, si rivolge alle famiglie con figli minori che non hanno diritto agli assegni familiari: ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, a quelle famiglie che non sono occupate da diverso tempo, alle famiglie indigenti. obiettivo condivisibile, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo e perché è imprescindibile il sostegno alla famiglia in maniera strutturale. modo, però, non sono più rinviabili i servizi a sostegno della natalità e gli incentivi alla promozione dell'occupazione prevalentemente femminile, perché effettivamente questa non è la misura a sostegno dell'occupazione femminile. *(Applausi)*. che il nostro Paese abbia il dovere di impegnarsi maggiormente per quanto concerne la spesa di protezione sociale per la funzione famiglia-figli, ben inferiore agli altri Paesi europei, con dati relativi al 2018 - lo voglio ricordare - distanti fra loro: circa l'1,1 per cento del PIL rispetto ad una media europea del 2,2 Tuttavia, il provvedimento in esame presenta alcune criticità, così come avevamo già rilevato, Ministro, in sede di discussione della legge delega sull'assegno universale e unico e le chiediamo davvero di tenerne conto nella stesura: molte famiglie ne sono escluse, a partire da quelle appartenenti al ceto medio, maggiormente bisognose di meccanismi di *welfare* per poter conciliare meglio vita e lavoro. Le risorse stanziate sono limitate: 3 miliardi per i prossimi sei mesi. Pertanto servono maggiori risorse per aumentare efficacemente la platea dei beneficiari. Ribadiamo anche in questa sede che per la determinazione dei destinatari si ricorre agli Indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), che però non garantiscono la massima copertura, perché pensiamo che oggi gli indicatori patrimoniali non sono più rispondenti alla reale situazione economica delle famiglie: si parte da una soglia minima di 7.000 euro fino ad una massima di 50.000 euro. Se, da un lato, questo sistema non incentiva ad aumentare il reddito (pensiamo per esempio ai percettori del reddito di

Sappiamo che la soglia dei 50.000 euro sarà facilmente oltrepassabile proprio per i patrimoni, che fanno parte della cultura del nostro Paese. Dal momento che questa misura si pone come intervento di sostegno alla famiglia, come ho già ricordato prima, ne sono interessati anche i percettori di reddito di cittadinanza. il problema non è tanto l'intervento di *welfare* rivolto anche a loro per la genitorialità, bensì il fatto che, com'è stato concepito - lo ripetiamo per l'ennesima volta - il reddito di cittadinanza non funziona *(Applausi)* e funzionerà ancora meno con l'aggiunta di ulteriori benefici. Simulazioni dell'INPS - lo voglio ricordare - prevedono entrate per i percettori di reddito di cittadinanza oltre i 1.150 euro mensili con tre figli a carico, quindi davvero un disincentivo al lavoro. Non si incentiva appunto l'occupazione, tantomeno quella femminile.

Il reddito di cittadinanza va dunque ripensato per trasformarlo finalmente da politiche passive a politiche attive. L'assegno temporaneo, così come l'assegno unico universale, è da intendersi come sostegno alla natalità e alla famiglia, non come sostegno al reddito. Forza Italia crede nel sostegno alla natalità, crede nel sostegno alla famiglia e al lavoro ed è per questo che, tra le proposte di riforma fiscale recentemente approvate nelle competenti Commissioni congiunte di Camera e Senato, Forza Italia ha inserito una detrazione fiscale importante per il secondo coniuge lavoratore, che in prevalenza è rappresentato appunto dalla donna. *(Applausi)*. In questo modo, oltre al sostegno economico per i figli a carico, viene incentivata l'occupazione femminile. Ritengo doveroso un cambio di passo anche in questo senso. Le misure degli ultimi anni hanno favorito l'assistenzialismo. Oggi questo assistenzialismo deve essere superato, in vista di una ripresa del sistema Paese, con interventi che stimolino le politiche attive per il lavoro. Di certo nessuno intende mettere in discussione la valenza sociale e morale degli aiuti per chi ne ha necessità, per chi è difficilmente inseribile nel mondo del lavoro, ma riteniamo che i sostegni debbano essere pensati per raggiungere degli obiettivi rispetto alla creazione di occupazione e di sostegno alla famiglia. Anche l'assegno ponte, però, non basta, così come non basterà l'assegno unico universale, che dovrà essere concepito come meno sostegno al reddito e più sostegno alla natalità, cui però non devono venir meno tutti i corollari per aiutare, soprattutto, le donne madri nel lavoro. Se si se si pensa al sostegno della genitorialità, non si può non pensare all'istituzione di un sistema integrato che preveda diversi servizi alla famiglia, tra cui gli asili nido, ad esempio, *(Applausi)*, il sostentamento economico, che deve essere tra l'altro equo per tutti. Se vogliamo raggiungere un livello di sviluppo pari ad altri Paesi europei, sfruttando le grandi opportunità del PNRR, dobbiamo necessariamente immaginare un sistema che si muove in maniera organica intorno alla famiglia, mettendo in connessione i diversi processi e non puntando esclusivamente all'assistenzialismo. In questo percorso che ci vede ripensare e modernizzare il sistema Paese lo Stato si deve porre in maniera diversa rispetto ai cittadini, deve assumere il ruolo di accompagnatore, anche per quanto riguarda la genitorialità. Le famiglie italiane sono la vera ricchezza e hanno bisogno di essere sostenute, di avere un lavoro per poter crescere i propri figli in serenità e questo è il vero sostegno: guardare ai figli significa guardare al futuro e dare valore al nostro Paese.

sappiamo perfettamente che l'argomento di oggi non è il tema definitivo. Ci stiamo occupando di un assegno ponte e, tuttavia, è bene ripartire dalle parole della senatrice Toffanin, che mi ha appena preceduto e che condivido in pieno, e cioè che dobbiamo affrontare la tematica della natalità con uno sguardo sistemico,

Mi faccio portavoce in questa Assemblea delle dichiarazioni dell'Associazione nazionale famiglie numerose, il cui presidente, l'amico Mario Sberna, che è stato parlamentare nella scorsa legislatura, ci ha messo in guardia dal fatto che l'assegno unico costituisca - parole sue - «una menzogna». Io non so se si arrivi a pensare questo, ma certamente i dati che Mario Sberna porta in quest'Aula meritano la nostra massima attenzione: secondo la ricerca dell'Associazione nazionale famiglie numerose, l'assegno unico non coprirà mai le detrazioni che verranno tolte e il meccanismo dell'ISEE va cambiato perché svantaggia le famiglie con più figli. Sempre secondo tale Associazione, metà delle famiglie numerose dovrà delle famiglie numerose dovrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, il che significa che questa norma è peggiorativa. Entriamo allora nel merito delle argomentazioni che i destinatari di questa norma pongono alla nostra attenzione. Ricordo ai colleghi in Aula che le famiglie numerose, cioè quelle con tre o più figli, sono le più esposte al rischio di scendere sotto la soglia di povertà: parliamo di un incremento,

di sostegno alla famiglia, cerchiamo almeno di farle bene, in modo che siano efficaci, che ottengano l'obiettivo e che non diventino mere norme di bandiera. Abbiamo tolto: gli assegni al nucleo familiare, le detrazioni per i figli a carico, le detrazioni per famiglie con quattro o più figli, l'assegno al terzo figlio, il *bonus* mamme, il *bonus* alla nascita. Tutto questo per dare in cambio un assegno unico, che tuttavia sarà parametrato in base al modulo ISEE. Io c'ero quando fu introdotto l'ISEE, quando fu realizzato questo iniquo sistema di calcolo delle sostanze familiari; c'ero e ricordo perfettamente chi era l'interlocutore che volle scrivere l'ISEE così come è scritto oggi, in maniera iniqua e ingiusta. Dobbiamo avere il coraggio di mettere mano all'ISEE e di trovare parametri che siano davvero confacenti a valutare i carichi familiari. Mi dovete spiegare che senso ha nel calcolo dell'ISEE introdurre la valutazione della quantità di denaro presente sul conto corrente al 31 dicembre. Sappiamo che le famiglie proprio in occasione del Natale ottengono regali, magari dai nonni o dagli zii, e li mettono sul conto corrente, e poi vengono penalizzate perché viene calcolato l'ISEE sulla base dell'ammontare del conto corrente al 31 dicembre. dicembre. Se avessero indicato il 25 del mese, anziché il 27 ad esempio, avremmo forse trovato il conto corrente vuoto perché appunto molte di queste famiglie non arrivano alla fine del mese. Al di là delle battute che purtroppo non sono tali ma realtà con le quali le nostre famiglie numerose stanno combattendo ogni giorno - noi abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto - e di questo ringrazio il relatore, che siede accanto a me

che per favorire le famiglie, che invece hanno diritto a una equa valutazione della loro ricchezza. Inoltre, come stavo dicendo, questa misura incide in modo molto pesante anche sulla situazione già molto delicata delle famiglie separate. Queste ultime e quelle che vivono la separazione e il divorzio vedono una ripartizione che, a nostro modo di vedere, è corretta e cioè: l'assegno unico viene erogato a metà tra i genitori che vivono la loro genitorialità nel regime di affido condiviso. Sappiamo che sono la stragrande maggioranza nel nostro Paese, oltre il 90 per cento; genitori meritano fiducia ed entrambi, partecipando alle spese di mantenimento e d'istruzione del figlio, meritano di ricevere, al 50 per cento di *default*, salvo ovviamente diverso accordo, l'assegno unico in pari misura. È altrettanto importante - e su questo abbiamo concordato - che l'assegno sia garantito e assicurato anche per coloro che non sono i genitori, ma che di fatto esercitano la responsabilità genitoriale sul minore. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Tuttavia, il piano culturale non può essere allontanato dal piano economico ed è su questo che vorrei concludere il mio intervento. La misura dell'assegno unico non risolve tutti i problemi, non è una panacea, non è la soluzione per venire incontro alle esigenze del nostro Paese in termini di natalità. Mi meraviglio nel leggere che l'assegno unico sarebbe la bacchetta magica, quando tutti noi sappiamo che portare un figlio dalla culla all'università costa circa 250.000 euro; ventiquattro anni significa 800 euro al mese. Se 800 euro al mese debbono essere pagati da ogni famiglia, ditemi voi, nella migliore delle ipotesi, quanto incide l'assegno unico: incide in una misura che non è neanche un quarto di ciò che le famiglie devono spendere per portare i loro figli all'università. Però vi faccio una domanda: una domanda: quei figli e quelle figlie, quando saranno laureati, a chi pagheranno le pensioni? A tutti noi che sediamo in quest'Aula, a tutti coloro che in questo momento stanno lavorando nel nostro Paese. Il fatto che i nostri figli e le nostre figlie possano arrivare alla laurea e a un lavoro che consenta loro di svolgere l'attività che preferiscono è o non è un bene per il Paese? Il fatto che di figli ne nascano tanti, che nascano i figli che ciascuna coppia desidera mettere al mondo è o non è un bene per il nostro Paese? Cominciamo a dirci queste cose, cominciamo a recuperare una cultura che si prenda cura delle famiglie che ogni giorno accompagnano i figli a scuola,

Noi stiamo dimenticando la famiglia e non sarà l'assegno unico a farcela ricordare. Servono politiche coraggiose. Serve togliere la voce famiglia dal capitolo spese per metterla sotto il capitolo investimenti.

Per il resto, c'è poco da aggiungere. Esprimo grande soddisfazione e ringraziamento alle colleghe, ai colleghi, alla Commissione al Governo. È stato fatto un lavoro veramente certosino. Ringrazio la Ministra per la pazienza con la quale ha saputo accompagnare

Il lavoro svolto ha visto nuovamente la trasversalità di tutte le forze politiche e credo che nuovamente si debba dare un riconoscimento estremamente positivo alla ricomposizione della politica che sui temi che riguardano l'educazione, le nuove generazioni, le famiglie e l'investimento in umanità sta mostrando l'immagine di un Paese coeso che sa finalmente operare scelte coraggiose e concrete.

assunto, per dare piena e pronta concretezza alla legge delega approvata dal Senato il 31 marzo e, dopo tre mesi, la possibilità di erogare già un assegno, seppure in una forma ponte, consegue esattamente a tale impegno. impegno. L'aver dovuto provvedere a una misura ponte corrisponde al fatto che l'annullamento delle detrazioni fiscali e degli assegni al nucleo familiare a metà anno avrebbe creato forti disagi alle famiglie. Abbiamo operato, anche in accordo con la Commissione, in piena coerenza con i principi della stessa legge delega. In realtà è un provvedimento di investimento nelle famiglie italiane. Le risorse dei 3 miliardi si aggiungono a tutte le altre risorse che già sono in essere. A nessuna famiglia italiana sarà tolto un euro: sono aggiunti

È un investimento e non un assistenzialismo. Sono d'accordo e condivido molto questa sollecitazione perché fa parte di una riforma. La misura al nostro esame è il primo pezzo di concretizzazione di un processo di riforma sistemica con l'assegno unico universale e che vede nel provvedimento del *family act* - tra l'altro proprio in questi giorni in discussione alla Camera - la piena realizzazione. Si tratta di un'integrazione di misure che riguardano l'educazione, il lavoro femminile, la condivisione dei carichi di cura e l'investimento sui giovani. Il tema della dimensione economica è certo importante. Rispetto ad alcune sollecitazioni avanzate rispetto anche alla quantificazione, purtroppo nel nostro Paese non siamo in una situazione di stato economico dei minori particolarmente vantaggioso. Secondo una recentissima simulazione dell'Istat, il 50 per cento dei minori del nostro Paese vive in nuclei familiari con meno di 10.000 euro di ISEE; ciò significa che al 50 per cento dei minori del nostro Paese arriverà un assegno compreso tra i

i minori esclusi, rilevo che i nuclei con più di 50.000 di ISEE sono circa il 3 per cento. Stiamo parlando di una misura universalistica proprio perché mantiene anche le detrazioni e perché ha una distribuzione anche di incidenza economica.

- e rispondono alla scelta di dare finalmente concretezza alle politiche di investimento per favorire la natalità, la genitorialità e l'educazione. Credo che ciò significhi dare al nostro Paese la piena attuazione delle pari opportunità per tutte e per tutti. Concludo con le parole del presidente Draghi, che ha citato gli stati generali della natalità, proprio parlando di questo strumento:

Per far sì che le nuove generazioni scelgano di avere fiducia nel loro futuro, il nostro compito è investire il nostro oggi nel futuro. E questo assegno è il primo passo di tale investimento.

dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge l'emendamento 6.0.1.

extraeuropei con figli minori a carico, ai quali non viene riconosciuto alcun assegno se privi dello *status* di rifugiato politico oppure di protezione internazionale. Lo sottopongo a voi tutti

Signor Presidente, con gli emendamenti 2.1, 2.4 e 2.0.1 sostanzialmente proponiamo delle alternative di calcolo rispetto

50.000 è una soglia che racchiude le categorie medie e, quindi, quelle famiglie in cui sono presenti due lavoratori che hanno uno stipendio medio.

tratta di una vera e propria modifica dell'ISEE: proponiamo la revisione del calcolo del reddito che oggi è al lordo delle trattenute; in questo caso lo proporremmo al netto delle accise regionali, comunali e anche

inversamente proporzionale al numero dei figli, e quindi più figli sono presenti nel nucleo familiare più si abbassa (5, 10, 15 e Proponiamo infine altri coefficienti in relazione alla presenza di anziani, di minori o di figli maggiorenni, lavoratori o meno, studenti o meno. Concludo dicendo che altra variazione di calcolo è il il coefficiente che dovrebbe stabilire le soglie ISEE, ed è una via di mezzo tra il quoziente familiare e il fattore famiglia.

del relatore. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.4, è stato dato un parere favorevole con una riformulazione sull'impegno al Governo. Si tratta di una modifica rispetto alla valutazione della situazione economica e reddituale di entrambi i genitori e non dell'ISEE:

è disponibile. Avendofatto la valutazione in Commissione, confermiamo la disponibilità.

Presidente, quella di oggi è una giornata importante, perché discutiamo di una norma che estende dei diritti, con conseguente arrivo di risorse alle persone che hanno più bisogno. Si introduce un assegno destinato alle famiglie con figli minori che finora non avevano diritto agli assegni al nucleo familiare. In particolare, l'assegno - come sappiamo - è diretto ai genitori disoccupati, lavoratori autonomi, precari o coltivatori diretti. Chiamiamo questo provvedimento ponte perché entra a regime dal 1° luglio al 31 dicembre, fino a quando il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico universale. In sostanza, mentre prima il sostegno della politica pubblica andava alle famiglie in ragione del lavoro o del non lavoro, e quindi della condizione dei genitori, ora l'assegno unico e universale sancisce un principio: l'aiuto è ai figli in quanto figli. È un cambiamento di dimensioni importantissime. In questo senso, la norma che ci accingiamo a votare è ponte, quindi, non solo perché stabilisce interventi immediati, ma anche prima avevamo isole separate, ossia ogni condizione di lavoro aveva il suo diritto all'assegno al nucleo familiare, mentre adesso il diritto è universale. in esame, però, è ponte anche verso la riforma più organica. Sono state richiamate riforme di sistema in quest'Aula, come il *family act*, approvato proprio l'altro ieri in Commissione affari sociali, che è una delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione delle famiglie e l'autonomia dei figli. Ringrazio la ministra Bonetti ed il Governo per un andamento ordinato delle norme, che consente di avere una visione più organica,

ad una fase almeno di convivenza e l'economia si sta riprendendo, tanto da far dire ad uno studio di Ambrosetti l'altro giorno che sta salendo il vento dell'ottimismo. questo vento dell'ottimismo deve spirare nella nostra cittadinanza, tra le famiglie, per innescare un processo di fiducia, di desiderio di futuro; fiducia che fa risollevare l'economia e l'occupazione e deve sostenere la natalità. Con alcuni colleghi, in modo trasversale ai partiti, abbiamo chiesto anche una sessione speciale del Senato del Senato sulla natalità, per affrontare il tema a tutto tondo. Tutto questo si accompagna alle riforme e alle risorse del PNRR. Ricordiamo che su queste tematiche sono appostate risorse importanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo ricordava la Ministra: ieri Draghi è tornato a parlare della condizione delle donne, appellandosi alle famiglie, è ora di agganciare questo tema alla ripresa economica. Draghi si è appellato alle famiglie e alle aziende, perché la la ricostruzione del Paese, a partire dal lavoro delle donne, ha bisogno di un investimento forte nel lavoro, nella parità di salario. questa la questione importantissima per affrontare il tema. In sostanza, la norma di cui discutiamo è una grandiosa leva di fiducia per il nostro prossimo futuro e per quello delle giovani generazioni.

ma con un misto di rabbia e di rincrescimento, interpretando anche il sentimento di tutte quelle famiglie nelle quali il Governo ha, incautamente, creato aspettative che sono andate deluse. Era tutto previsto e potremmo riprendere gli atti della seduta del 30 marzo scorso, nella quale abbiamo approvato all'unanimità la misura dell'assegno unico universale per i figli, e quindi con il voto favorevole anche di Fratelli d'Italia, come accaduto anche alla Camera otto mesi prima. Già il 30 marzo, però, abbiamo stigmatizzato il ritardo e i tempi stretti di una riforma che sarebbe dovuta entrare in vigore il primo luglio e che sconta un errore all'origine, nella vostra scelta di un disegno di legge delega, i cui tempi sono sempre incerti e lunghi. Era già evidente che non c'erano gli spazi sufficienti per varare i decreti attuativi, che sono gli unici deputati a garantire una copertura adeguata e l'entrata in vigore della misura. D'altronde - e non è casuale - il Governo non era in grado di quantificare la cifra dell'assegno e gli interventi del Ministro di competenza, ma anche del Presidente del Consiglio, si basavano su previsioni e simulazioni che oggi potremmo definire con il loro nome, e cioè campate per aria. Infatti, si è ricorso a una soluzione ponte, da luglio a dicembre: l'assegno temporaneo. Ad aprile era già evidente che l'assegno unico era condannato a rinvio, ma solo con ritardo è stata ufficializzata la misura che oggi discutiamo. Insomma, il Governo ha nascosto le strettoie legislative e burocratiche, che pure conosceva. Sta vendendo come vittoria l'assegno temporaneo, che invece è un insuccesso politico. Il piano B del Governo, la soluzione ponte, permette di salvare il salvabile grazie ai tre miliardi aggiuntivi stanziati nella finanziaria 2021, ma non bastano. Inoltre, siamo lontanissimi non solo dalla filosofia del *family act*, ma proprio dal principio della universalità dell'assegno unico, che dovrebbe appunto riguardare tutti e riunire, in una sola misura, le misure oggi esistenti. Si tratta di circa sei sussidi diversi. Insomma, con una battuta direi che per il il Governo vale il principio di università quando si tratta di dare monopattini a tutti; ma, quando si tratta di pagare i pannolini per i neonati, improvvisamente si abbandona l'universalità e si diventa restrittivi. *(Applausi)*. Si vorrebbe introdurre un cambio di paradigma nelle politiche di sostegno alla famiglia, della natalità e della demografia e, invece, oggi si concretizza una sorta di ulteriore *bonus*, sganciato da una visione

di un corto circuito legato alla certificazione dell'ISEE, che è uno strumento iniquo e discriminatorio, che Fratelli d'Italia ha proposto di modificare, come hanno già spiegato i miei colleghi, senatori Maffoni e Drago, che ringrazio per il lavoro svolto. L'ISEE è molto distante dal principio dell'universalità come dell'equità e, soprattutto, è distante da un'etica di inclusione, che è meglio rappresentata - a nostro avviso - dall'idea di quoziente familiare e dal modello di fattore famiglia. famiglia. Ricapitolando, al di là delle dichiarazioni trionfalistiche, la verità è una: il Governo è rimasto impantanato sull'assegno unico e il suo *storytelling* prevedeva che la misura entrasse in vigore il 1° gennaio 2021, poi è scivolata al 1° luglio. In realtà, la legge delega entrerà in vigore - speriamo - nel gennaio 2022,

Si è fatta della demagogia; si è nascosto fino all'ultimo lo slittamento dell'assegno unico al 2022. D'altronde, i soldi non c'erano; quelli stanziati erano insufficienti; quelli del *recovery* ancora non ci sono e l'assegno unico e universale è inserito nelle riforme di accompagnamento al Piano nazionale di ripresa

cari colleghi, è che nessuno avrà mai i 250 euro promessi. *(Applausi)*. Infatti, si va da un minimo di 30 euro a un massimo di 217 euro mensili per figlio e l'importo dell'assegno in base al ISEE cala, per poi crollare, per chi supera i 50.000 euro. stiamo parlando di un *bonus* temporaneo che riguarda una platea ristretta di famiglie, quelle che non godono degli assegni familiari. Stiamo parlando di 2 milioni di persone, tra lavoratori autonomi, disoccupati, incapienti, inattivi, lavoratori dipendenti esclusi per ragioni di reddito dagli assegni familiari; per non parlare della logica perversa dell'accumulo con il reddito di cittadinanza, quello che aveva abolito la

che infatti sono le grandi assenti del PNRR, e nessuna delle sei missioni è dedicata in modo specifico - come invece ha richiesto Fratelli d'Italia - alla famiglia e alla natalità. Al Governo sfugge evidentemente quanto costa un figlio, e non lo dico io, ma lo dicono gli studi di politica economica: costa tra i 250 e i 350 euro

In sintesi, la nostra mozione chiede che il Governo rispetti almeno i tempi previsti e gli impegni assunti per la data di decorrenza del gennaio 2022, introducendo il fatidico, famoso assegno unico e soprattutto eviti che le famiglie vadano, al netto, a percepire di meno di quello che percepiscono oggi. È stato fatto un calcolo, e lo voglio dire: due milioni di famiglie, cioè il 22 per cento della platea, rischiano con l'assegno unico, quello futuribile, di andare a prendere di meno e sto parlando in particolare delle famiglie numerose. Torniamo all'assegno temporaneo, che è individuato in base ai livelli di ISEE e ha degli importi bassissimi per il ceto medio e comporta il rischio - lo sottolineo, Presidente - di una vera e propria trappola della povertà

dovesse esprimere un giudizio sull'operato del Governo su questa materia, noi dovremmo votare due volte contro, ma Fratelli d'Italia ha nel suo DNA di valore, nonché nei suoi programmi in sostegno alla natalità e alla famiglia, combattere il *trend* demografico negativo. È solo con questo spirito, quello di un'opposizione responsabile, che come in precedenza esprimiamo un sofferto voto favorevole a questo provvedimento. Lo facciamo per quelle famiglie, in quella logica tristanzuola del «piuttosto di niente è meglio piuttosto». Ma un Governo che strombazza come fatto addirittura epocale uno straccio di assegno temporaneo si assuma la responsabilità di essere venuto meno a una promessa, e deve essere consapevole che le famiglie non vogliono regali, ma giustizia sociale e riconoscimento del loro ruolo.

il decreto-legge che stiamo per convertire contiene una misura di grande importanza: l'assegno temporaneo per i figli minori, che è l'assegno ponte nelle more della riforma dell'assegno unico e universale per le famiglie che abbiamo approvato con la legge delega n. 46 di quest'anno: una legge delega importante, che ha visto il coinvolgimento e il protagonismo di molti attori politici; una legge delega di origine parlamentare, proposta dal Partito Democratico sia alla Camera sia al Senato, sulla quale

Ricordo la cornice solo per sottolineare che l'assegno temporaneo si chiama sì temporaneo, ma non è un *bonus* tra tanti e non è un *bonus* passeggero: è l'anticipo e il trampolino verso una riforma di sistema che dovrà rendere il nostro fisco e i trasferimenti monetari del nostro *welfare* più forti e generosi nel sostenere natalità e genitorialità. una riforma importante per contrastare l'inverno demografico in cui il nostro Paese è calato da decenni. Non c'è una statistica economica del mercato del lavoro o della sostenibilità del *welfare* che non sia imputabile in chiave negativa a tale inverno demografico, per questo abbiamo bisogno di un fisco e di un *welfare* più generosi per le famiglie con figli. È una riforma importante anche per superare le iniquità del sistema precedente, soprattutto quelle orizzontali e verticali rispetto ad alcune categorie, a partire da lavoratrici e lavoratori autonomi e incapienti. È anche importante che questa riforma - lo sottolineo di nuovo - sia stata votata all'unanimità, perché questo mette al riparo le misure di contrasto all'inverno demografico dall'instabilità politica e dalla volatilità delle maggioranze parlamentari di turno. È quanto avvenuto in altri Paesi come la Francia, dove politiche di svolta e di contrasto al declino demografico sono state portate avanti grazie all'accordo di tutte le forze politiche. Proprio perché l'assegno unico e universale è una riforma di sistema, era ed è necessario farla bene e con i tempi giusti. Quindi è bene che parta dal 2022, ma era altresì necessario usare le risorse del 2021 e dare subito un segnale di intervento. Per questo mi associo al ringraziamento e all'apprezzamento per il lavoro su questo provvedimento svolto dal Governo, dalla ministra Bonetti e dal Parlamento, a partire dal relatore, il collega Laus, e dalla presidente Matrisciano. Negli stretti vincoli temporali e finanziari in cui si muoveva questo intervento, si è fatto il possibile per usare le risorse del 2021 partendo da due platee, autonomi e incapienti, che erano anche quelle svantaggiate dal sistema precedente. È stata la scelta giusta, ma ora ogni sforzo deve concentrarsi sull'assegno unico e universale a regime, di cui l'assegno temporaneo rappresenta un ponte, ma non deve rappresentare una fotocopia. Ci sono molti nodi ancora da sciogliere e non era possibile farlo, con questi tempi e con queste risorse, ma andrà fatto con i decreti legislativi, spiegando a maggior ragione che l'assegno temporaneo è soltanto un ponte verso qualcosa di diverso per non generare aspettative acquisite a cui non saremo in grado di rispondere. I nodi a mio avviso sono soprattutto due. Innanzitutto, ribadire l'universalità dell'intervento. Universale non deve essere solo l'aggettivo del nome dell'assegno a regime, ma deve essere la cifra della filosofia della misura che vedrà la luce nel 2022. Un universalismo selettivo, giustamente, ma con una selettività temperata, che faccia capire che l'assegno unico e universale non è una misura di contrasto alla povertà

pezzo ampio e generalizzato della popolazione italiana e dei ceti medi. Questo è il primo nodo da sciogliere. Il secondo nodo riguarda l'occupazione femminile. fare in modo che a regime l'assegno non scoraggi l'occupazione femminile. Sappiamo che i trasferimenti monetari portano sempre con sé un disincentivo all'offerta di lavoro, soprattutto di chi ha redditi bassi - e purtroppo in Italia questo

Questi due obiettivi hanno bisogno di sciogliere due questioni: come usiamo l'ISEE nell'assegno unico universale e se le risorse che abbiamo a disposizione sono sufficienti o hanno bisogno di un *pit stop* con la legge di bilancio. Sull'ISEE penso che dovremmo usare tutti i gradi di flessibilità che la legge delega contiene sull'impiego delle sottocomponenti, per ridurre l'eccessiva progressività dell'assegno temporaneo, per attenuare alcuni vincoli patrimoniali, che potrebbero lasciare fuori una parte dei ceti medi, e per rendere la misura veramente giorno, accolto dal Governo - ragionare su come rendere meno forte il peso del reddito del secondo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare per favorirne l'occupazione, dato che in molti casi ancora vuol dire occupazione femminile. Il secondo nodo sono le risorse: dobbiamo capire se sono sufficienti. Probabilmente, se vogliamo fare una misura veramente universale e ridurre la progressività eccessiva dell'assegno ponte, abbiamo bisogno di altre risorse. Abbiamo bisogno di almeno due miliardi di l'assegno unico e universale non raggiunga solo autonomi e incapienti, ma dia una risposta vera anche al lavoro dipendente e ai ceti medi. L'ultimo punto - e chiudo - è che, come ricordava la collega Fedeli, l'assegno unico e universale rappresenta una riforma importante solo e fintanto che è inserita in una strategia complessiva di sostegno alla genitorialità, alla natalità

valorizzare per realizzare una rete forte di servizi educativi destinati all'infanzia e al sostegno alla genitorialità. passare da politiche di conciliazione a politiche di condivisione, affinché la scelta di andare incontro al desiderio di avere figli,

politiche di condivisione. Per questi motivi e dentro questa cornice, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico su questa importante

mi unisco anch'io ai ringraziamenti che sono stati ampiamente formulati dai colleghi che mi hanno preceduto verso il relatore, senatore Laus, la Presidente della Commissione, e la

che delega il Governo a costruire lo strumento dell'assegno unico che abbiamo votato in quest'Aula, su cui abbiamo ampiamente dibattuto e su cui torneremo naturalmente in fase di implementazione. È un provvedimento importante in sé perché rappresenta una sorta di *stress test* proprio in vista del percorso di implementazione di quella riforma,

ha ragione chi mi ha preceduto: è difficile dividere il giudizio e la valutazione sul provvedimento, che abbiamo definito ponte, temporaneo, dalla valutazione complessiva del processo di riforma di cui stiamo parlando. In questo senso faccio tre brevissime considerazioni. In primo si è parlato di un tratto che io penso debba informare l'intera cornice delle politiche di *welfare* che mettiamo in campo, cioè quello universalistico. Con il provvedimento al nostro esame diamo un contributo ad aumentare di qualche grado proprio il tratto di universalismo degli strumenti che oggi sono presenti e che sono a nostra disposizione, perché l'assegno temporaneo amplia la platea dei beneficiari, includendo categorie che altrimenti non sarebbero state destinatarie di una misura così importante. Penso ai lavoratori autonomi, ai disoccupati

trascurato dal punto di vista di un'attenzione che invece andava tenuta alta e che oggi non possiamo più non porre, tanto più alla luce di quello che è accaduto in questi mesi. Abbiamo scoperto una cosa che avremmo dovuto sapere già prima,

neo proletariato. Rischiamo cioè di misurarci con persone che, nonostante il lavoro che naturalmente hanno messo in campo con la ragione del proprio talento, non riescono a sostenere se stesse e i propri cari e, quindi, a far sì che quel lavoro produca un salario dignitoso. Stiamo parlando di una difficoltà vera, reale, di condizioni materiali, di persone che abbiamo scoperto in pandemia molto più fragili di quanto non immaginavamo. Da questo punto di vista aumentare l'universalità di strumenti come quelli che stiamo mettendo in campo, includendo anche categorie di questo genere, va nella direzione giusta, disegna la prospettiva di un mondo del lavoro non segmentato, dove non ci sono lavoratori di serie A o di serie B, lavoratori che godono di sistemi di protezione e quelli che non

e dentro quella famiglia realizzare il sogno di avere dei figli e di mantenerli materialmente. Con questo tema ci dobbiamo misurare. Da questo punto di vista, punto di vista, l'assegno temporaneo e l'assegno unico che verrà costruito rappresentano un elemento molto importante - hanno ragione alcuni colleghi che mi hanno preceduto - solo a patto che siano un pezzo di una strategia complessiva. Lo diceva molto bene la collega Fedeli in discussione generale. Dobbiamo ragionare in termini di sistema e non dobbiamo innamorarci di formule che sono molto affascinanti nella loro proiezione pubblica, ma che, quando vengono precipitati nella loro implementazione, risolvono molto poco dei problemi che sollevano.

la condizione materiale delle persone dipende anche dal *set* di beni pubblici che lo Stato è in grado di garantire alle donne e agli uomini. Quel pezzo che si aggiunge al reddito che quelle donne e quegli uomini riescono a produrre con il loro lavoro fa effettivamente la differenza. È un fatto di condizioni materiali, ma anche di possibilità di continuare a svolgere la propria esistenza con dignità. Infine, ci sono le criticità; le ha sottolineate anche il relatore nella sua sua relazione. Non entro negli aspetti più tecnici perché ci sarebbe molto da parlarne. C'è un elemento di accentuazione della misura per famiglie con almeno tre figli. Presidente, Presidente, per il suo tramite lo dico al senatore Pillon: in questo caso non c'è il tema che lui sottolineava; semmai c'è il tema contrario, che deriva dal fatto che non si capisce perché non si debba ammettere che ci siano effettivamente economie di scala - scusate l'espressione - tra avere una famiglia con due figli e averne una con tre. Quel rapporto in qualche modo andrà regolato, altrimenti non si capisce se la misura è pronatalista o se effettivamente si occupa del fatto che le famiglie più numerose siano più a rischio povertà. In ogni caso,

sola battuta con l'unica nota polemica del mio intervento: smettiamola di attaccare il reddito di cittadinanza e, soprattutto, di costruire una correlazione che non esiste che non è significativa tra le misure di sostegno al reddito e il presunto disincentivo che queste misure creerebbero alla ricerca del posto del lavoro. Non c'è nessuno in questo Paese che vuole poltrire sul divano aspettando un sussidio pubblico. Semmai ci sono donne e uomini che vogliono avere un lavoro dignitoso, e per trovare i lavoratori che non si trovano - mettiamo da parte anche questa discussione pubblica molto stucchevole - basta pagarli di più e

e l'assegno temporaneo, perché questo ha un impatto sulle dinamiche di risparmio delle famiglie e sull'impianto progressivo generale. Ripeto, è una questione tecnica che però ha una sua importanza, che verrà e dovrà essere attenzionata quando dovremo occuparci della fase implementativa dell'assegno unico. Per queste ragioni, e anche alla luce delle criticità che ho sottolineato, voteremo a favore del provvedimento e naturalmente ci impegniamo a migliorare il percorso di strutturazione dell'assegno unico quando ne avremo - molto presto - l'occasione. Signor Presidente, signora Ministro, colleghe e colleghi, non replico - per rispetto delle opinioni - all'intervento che mi ha preceduto, ma svolgo il mio intervento così come avevo previsto. Come avevamo segnalato durante l'esame della legge delega sull'assegno unico per i figli, anche con questo decreto-legge sono emerse diverse criticità e iniquità. Rimane comunque la nostra volontà di votare a favore del provvedimento, nella considerazione che le risorse a favore delle famiglie aumentano per ulteriori 3 miliardi, anche se non avviene nel modo e nell'ammontare che avremmo voluto. Soprattutto è apprezzabile il fatto che a percepire l'assegno saranno, per la prima volta, anche i lavoratori autonomi e persino i disoccupati. Di negativo resta il fatto che l'assegno sia ancora legato a parametri che non fotografano l'esatta situazione reddituale e patrimoniale di una famiglia, con un meccanismo troppo selettivo che decresce troppo velocemente. Rileviamo poi il problema ulteriore delle famiglie sposate, che sono di fatto discriminate rispetto a quelle non sposate. La somma del reddito di due persone sposate fa registrare un ISEE più elevato rispetto a quello di due persone che convivono. L'assegno per due persone che convivono sicuramente verrà richiesto dal *partner* con il reddito più basso, per cui non c'è cumulo di reddito in questo caso. Ancora, la procedura prevede che tutti coloro che vogliono l'assegno devono richiederlo all'INPS, come se lo Stato non fosse già a conoscenza di chi ha figli e di quanti ne ha. La richiesta invece non deve essere presentata dai percettori del reddito di cittadinanza, che uniranno ora un assegno al reddito pubblico, non preoccupandosi la norma della rioccupabilità di questi padri di famiglia che nella loro dignità avrebbero dovuto cercare di essere invogliati a trovare un lavoro anziché un reddito che peraltro non li arricchirà sicuramente. Insomma, è una riforma che discrimina chi ha reddito superiore a 50.000, cioè circa 2.300 euro al mese - questa è la cifra di cui parliamo - che non penso possa essere discriminato in quanto tale, ma soprattutto disincentiva la creazione della famiglia classica, quella sposata con figli, come l'abbiamo sempre conosciuta. Questo assegno deve essere quindi solo un passaggio temporaneo - per questo voteremo a favore - che dovrà essere modificato da una riforma complessiva dell'intero sistema fiscale disegnato a misura della famiglia, come già chiesto nella riforma fiscale da Forza Italia. contrario, si rischia di creare uno Stato meramente assistenzialista, che è forse l'obiettivo di alcune presenze in quest'Assemblea. Lasciatemelo dire con una battuta: se persino uno Stato comunista come la Cina ha abbandonato la politica del figlio unico per passare all'incentivo ai tre figli, con la politica dell'assegno unico rischiamo di andare verso un modello persino peggiore di quello comunista. Il modello può essere per noi quello tedesco, dove l'assegno ai figli non ha livello di selettività, ma soprattutto possiede il carattere dell'universalità. Ma può essere anche quello francese, dove è previsto il quoziente familiare, in cui la riduzione non è così drastica come quella italiana; 7.000 euro si prende tutto, poi si arriva a risorse intorno ai 30.000-35.000 euro l'anno di ISEE, che rappresentano veramente uno stipendio che non arriva a 2.000 euro al mese. Un'imposta,

dove la differenza non la fa l'assegno per il figlio o meno, ma il reddito che rimane a disposizione della famiglia, al netto di tutte le tasse che gravano sul nucleo familiare, comprese quelle sulla casa. Inoltre, noi pensiamo che anche l'accesso alle strutture che provvedono alla crescita e alla formazione dei nostri ragazzi, come gli istituti, le scuole e le università, debba essere agevolato per tutti e non legato al reddito; deve essere reintrodotto anche il merito. Un tempo gli studenti che avevano un buon profitto avevano l'esenzione dalle tasse,

sono veramente meritevoli le borse di studio se le vanno a prendere all'estero, dove le danno agli studenti meritevoli; con la differenza che lì rimangono, lì lavorano e lì mettono a frutto le loro capacità.

Non dobbiamo punire le famiglie monoreddito, in cui uno dei genitori ha scelto di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. Anche noi siamo ovviamente a favore della piena occupabilità femminile; ma, in assenza di un lavoro, il fatto di occuparsi dei figli a tempo pieno deve avere un pieno riconoscimento sociale ed economico, in attesa di vedere tutte le mamme inserite nel mondo del lavoro. Invece non c'è alcun premio per chi si prende cura direttamente della famiglia e non scarica questi oneri sulla società e sul nostro *welfare*. A noi adesso sembrano mal coniugate le ragioni di favorire le donne che lavorano con quelle che invece danno il giusto sostegno economico alle mamme; ma non ci deve essere contrapposizione tra la donna che lavora e la donna che sta a casa, in attesa di vedere

avendo tutte le strutture sociali che consentano questo (la scuola che dura fino alle 16, il tempo pieno, gli asili nido). Ma questo è un argomento che affronteremo nel prossimo futuro. Si dovrebbero quindi attivare anche le agevolazioni sulla genitorialità, che mancano in questo provvedimento e che però sono previste dalla legge delega che abbiamo approvato e che speriamo di dover riesaminare a breve.

In definitiva, fatte le puntualizzazioni che ho appena espresso e sicuramente altre considerazioni che a breve riprenderemo, i senatori

una senatrice che con tenacia ha difeso un concetto imprescindibile per noi della Lega: prima gli italiani, prima le politiche attive del lavoro

Ci tenevo a dirlo in maniera ufficiale e davanti a tutto il Gruppo, perché sei un esempio. Stavo ascoltando alcuni interventi riguardanti il reddito di cittadinanza (ho preso degli appunti al volo) volo) e anche la compressione degli stipendi dei lavoratori italiani, però dobbiamo anche chiederci per quale motivo i lavoratori italiani hanno perso diritti: forse a causa delle privatizzazioni targate Prodi, Bersani, Letta,

del contratto collettivo nazionale e delle parti sociali? Io porto sempre l'esempio della famosa società Groundcare, un'azienda dell'aeroporto di Fiumicino, ex ADR trasformata in Groundcare e poi successivamente subappaltata a un'azienda straniera.

Anche Alitalia e Telecom hanno subito questa depressione sociale, desidero chiamarla così. Venendo al provvedimento che ci accingiamo ad approvare, il decreto-legge in esame ha una durata di sei mesi, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. La Lega, proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli, lo sostiene con forza, perché la famiglia è una istituzione fondamentale per la tenuta sociale della Nazione. Rafforzare le politiche per tutelare la famiglia è fondamentale; ovviamente parlo della famiglia biologica, non dei modelli sintetici creati in laboratorio o delle teorie fluide per assecondare i capricci La famiglia biologica è importante per la sopravvivenza di una Nazione e a causa della crisi economica moltissimi nuclei familiari vivono momenti difficili. Per questo è importante dare delle risposte. Il decreto-legge è un provvedimento ponte, ma anche nel merito l'assegno familiare è un passo importante; tuttavia l'obiettivo finale della Lega è il quoziente familiare e più in generale la *flat tax,* una tassa piatta che terrebbe conto dei carichi familiari per individuare alcune zone *no flat tax.* Come ha detto

colleghe e colleghi, siamo chiamati oggi a convertire in legge il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che reca misure temporanee e provvisorie in attesa dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla legge del 1° aprile 2021 n. 46. È una legge relativa al riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale. È una riforma, quella di cui alla legge delega, di fondamentale importanza per tutte le famiglie di questo Paese ed entrerà a regime da gennaio dell'anno prossimo. È un intervento importante perché con il decreto-legge in conversione intendiamo anticipare temporaneamente gli effetti di questa legge; li estendiamo ai nuclei familiari che in ragione dei profili soggettivi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'assegno per il nucleo familiare che è vigente oggi. Parliamo di un passo in avanti per tutte le politiche di *welfare* di questo Paese, che avvicina l'Italia all'Europa e che per la prima volta estende gli aiuti previsti per i lavoratori dipendenti con i figli per i quali il provvedimento in questione interviene, prevedendo una maggiorazione per ciascun figlio, anche a categorie che fino ad oggi sono rimaste escluse come ad esempio i lavoratori autonomi. Grazie al lavoro nelle Commissioni di merito, sono state infatti apportate delle modifiche migliorative al testo che è stato licenziato dal Governo e che oggi è all'esame dell'Assemblea; mi riferisco in particolare alla Commissione lavoro del Senato, che ha esaminato l'assegno temporaneo in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre regime, quando entrerà a regime la riforma e lascerà quindi il posto all'assegno unico universale, come voluto dal Governo Conte II, dal MoVimento 5 Stelle e dall'ex ministra Nunzia Catalfo. Una tra tutte è quella modifica che punta a promuovere l'effettiva parità tra i generi, stabilendo che l'assegno temporaneo venga corrisposto dall'INPS e ripartito in misura pari tra i genitori, ad eccezione di alcuni casi particolari espressamente citati dalla norma. È un segnale importante, a nostro avviso, in questo momento complesso perché segnato dalla pandemia e che rimarca la necessità di assicurare pari condizioni ed opportunità a uomini e donne, nel rispetto dei principi costituzionali e soprattutto nel rispetto di quel principio di effettiva uguaglianza sostanziale tra i sessi e più in generale delle persone, intese con la P maiuscola. In un Paese con un basso tasso di natalità, incentivare la genitorialità, sostenere la famiglia con aiuti economici concreti per ciascun figlio a carico o un nuovo nato è certamente importante, soprattutto se guardiamo ai nostri giovani e ai precari, troppo spesso costretti a rinunciare alla gioia di diventare genitori perché magari non hanno un lavoro stabile che sia in grado di assicurare a loro stessi e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questo decreto ponte è una misura temporanea e il prossimo *step* sarà quello di dare piena attuazione alla riforma che, nell'introdurre l'assegno unico universale, prevede una razionalizzazione di quei micro aiuti che sono previsti per chi ha figli e che dalle leggi vigenti sono spesso frammentati e necessiterebbero di lungaggini burocratiche e diversi passaggi prima di arrivare nella disponibilità dei cittadini. Da gennaio 2022, invece, le famiglie italiane, a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai ventuno anni per ciascun figlio a carico, potranno finalmente contare su un assegno unico e universale che rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese. Lo Stato ha il dovere di abbattere le disuguaglianze e sostenere i cittadini, promuovere pari opportunità per tutti e con questo strumento compiamo un ulteriore passo in avanti anche a tutela delle nuove generazioni. Per questo motivo, esprimo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, il disegno di legge costituzionale sarà approvato, in sede di seconda deliberazione, se nella votazione finale otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

deliberazione di un disegno di legge di riforma costituzionale molto importante, già esaminato dall'Assemblea del Senato nel settembre 2020 e che affronta oggi il suo quarto passaggio parlamentare. Ricordo che il 31 luglio 2019 c'è stata la prima lettura alla Camera, il 9 settembre del 2020, come ricordavo, la seconda lettura del Senato e lo scorso 9 giugno la seconda deliberazione della Camera dei deputati. In tutte queste votazioni c'è stata un'adesione molto ampia dell'Assemblea parlamentare in favore di questo provvedimento che, come si sa, è davvero semplice nella sua natura. Si tratta di una modifica dell'articolo 58 della Costituzione, al primo comma, fatta per consentire che si abbiano elettorati uguali per l'elezione di entrambi i rami del Parlamento, in modo che i diciottenni possano eleggere anche la Camera alta. È una modifica che si traduce nella eliminazione, dal comma 1 dell'articolo 58 della Costituzione, di dieci parole; ma è una modifica che, togliendo dieci parole, opera in realtà un grande cambiamento, perché rimuove, dal nostro sistema istituzionale, un'anomalia che da lunghissimo tempo si tentava di eliminare e che non si è riusciti a eliminare, nonostante molti tentativi e discussioni. A me fa piacere ricordare che dell'equiparazione degli elettorati per l'elezione dei due rami del Parlamento si discute, nel dibattito pubblico italiano, perlomeno da quando, nel marzo del 1975, quindi tantissimi anni fa, venne approvata la legge di riforma del diritto di famiglia, con l'abbassamento da ventuno a diciotto anni della maggiore età. necessario a vasti settori della politica italiana, anche per il mutare dei tempi e dei costumi, superare la diversificazione degli elettorati delle due Camere, per una ragione sia funzionale sia di equità intergenerazionale. non ci si è riusciti. Ricordo, tra i tanti tentativi, un disegno di legge costituzionale, anticipatore e molto lucido soprattutto nei contenuti della sua relazione, presentato nel luglio del 1987 dal senatore Mancino, che poi sarebbe diventato, nella XIII legislatura, Presidente molto apprezzato di questa Assemblea. Adesso siamo davvero ad un passo dal traguardo e ci sono tutte le condizioni perché, anche al Senato, nella seconda deliberazione si possa arrivare ad un voto favorevole ampio in favore di questo provvedimento. Ricordo soltanto che con l'approvazione di questo provvedimento facciamo in modo che che quattro milioni di italiani escano dalla situazione di minorità e di inferiorità civile nella quale si trovano oggi, perché esclusi dal diritto di votare una Camera che esercita, su un piede di perfetta parità con l'altra, il potere legislativo: una differenziazione che, come dicevamo prima, non ha davvero più alcuna ragione d'essere. Oltre a questa ragione di equità, c'è una motivazione di funzionalità, perché sappiamo che avere elettorati uguali per le due Camere abbassa, fin quasi ad azzerare, uno dei rischi che molte volte ha costituito un problema per il funzionamento ordinato delle nostre istituzioni, cioè quello di maggioranze diverse nelle due Camere in conseguenza di elettorati differenti. ho creduto fosse necessario accompagnare ad una relazione puramente descrittiva di una modifica, che quantitativamente è poca cosa, anche un ricordo dei motivi essenziali di natura politica e costituzionale che rendono questo provvedimento estremamente importante. Dopo aver importante. Dopo aver approvato a larghissima maggioranza la riforma che introduce la tutela ambientale in Costituzione, abbiamo nell'Aula del Senato una nuova occasione di scrivere una buona pagina di riformismo costituzionale.

con finalità non ostruzionistiche, ma assolutamente collaborative, una soluzione che vada bene a tutti: ad esempio, un'interruzione alle 18,30 o la garanzia che il voto una parte delle dichiarazioni di voto si possa svolgere domani mattina. Quindi, chiedo a lei di trovare un punto di equilibrio. A noi interessa poter svolgere la nostra riunione di Gruppo al massimo entro le 18,30. Questa è la nostra richiesta. Signor Presidente, ovviamente aderiamo alla richiesta del presidente Ciriani. Lo avevamo già fatto, ma semplicemente per un *misunderstanding* non ci siamo coordinati sugli orari.

Presidente, non siamo d'accordo sul chiudere alle 18,30. Se i colleghi vogliono fare la riunione di Gruppo, noi siamo per proseguire la discussione generale, anche perché poi abbiamo la richiesta - come ho già preannunciato ai colleghi - di modifica

Abbiamo cinque interventi in discussione generale, quindi alle ore 18,55 avremmo concluso svolgere la discussione generale, interrompere la seduta a quel punto e lasciare le dichiarazioni di voto e il voto finale per la giornata di domani mattina. Può essere una proposta accoglibile, senatore Ciriani?

non mi pare dignitoso per l'ultima lettura di una riforma costituzionale. Questa è la mia opinione.

certo, che orientativamente dovrebbe essere domani mattina alle ore 11. In questo modo, si potrebbe garantire quella maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione.

dei nostri Padri costituenti. Ho il dovere, da cittadino di questa Repubblica, da persona che ha studiato all'università e che crede nelle istituzioni, di dire che questo sistema di modificare la nostra Costituzione

l'umile ultimo dei 315 senatori che seggono qui. Lo dicono Presidenti della Corte costituzionale, costituzionalisti, persone - badate

a fare le riforme costituzionali è sbagliato. *(Applausi)*. Non è così che si modifica la nostra Costituzione.

del voto ai diciottenni (che non gliene può fregare di meno, perché in questo momento i diciottenni pensano a tutt'altro che a votare anche per il Senato oltre che per la Camera dei deputati), ma non ci stiamo minimamente preoccupando di quel che dovremmo fare, avendo ridotto di quasi il 40 per cento il numero Se non ci sbrighiamo, probabilmente saremo costretti ad affrontare le prossime elezioni politiche con una serie di caducità, di problematiche, di questioni non solo regolamentari, ma anche costituzionali, che non consentiranno a queste due Camere di funzionare. Ho depositato, con la firma di molti miei colleghi, a cominciare dalla presidente del mio Gruppo Anna Maria Bernini, un disegno di legge costituzionale che tenta faticosamente di mettere una pezza ai problemi che purtroppo scaturiranno da questo populistico e incomprensibilmente drastico ridimensionamento del numero dei parlamentari della nostra Repubblica. Ma veniamo alla questione del voto ai diciottenni.

Se la Camera e il Senato devono avere, anche dopo la riduzione dei parlamentari, un numero differente di componenti (perché da una parte saranno saranno 400 e dall'altra 200), allora mi si deve spiegare perché dovremmo adeguarlo in tutto. Allora dovremmo adeguarlo anche nel numero dei parlamentari? Ascoltai questa affermazione dal presidente Calderoli in 1a Commissione affari costituzionali e lo applaudii, non c'è coerenza tra la riduzione dei parlamentari, l'adeguamento, perfettamente identico, tra Camera e Senato e poi - chissà perché - un numero differente di membri nell'una e nell'altra Camera.

nel quale sia comprensibile a cosa deve servire la Camera dei deputati e a cosa deve servire il Senato della Repubblica. Altrimenti, se noi non spieghiamo questo, non basta dire: diamo un segnale ai diciottenni, a quelli che ce l'hanno con la politica, la politica, a quelli che pensano che i parlamentari rubino lo stipendio, per cui è meglio ridurre il numero dei ladri di stipendi. Tutto questo non ha alcun senso, è solo frutto di un'assurda mentalità antipolitica, che non fa riconquistare fiducia ai cittadini nelle istituzioni, anzi, contribuisce a farla perdere. Perché guardo con speranza alla Presidenza Draghi? Perché finalmente abbiamo una figura autorevole, che non pensa a dare segnali populistici, a *spot*, per cercare di conquistare il consenso, ma cerca soltanto di dare una prospettiva e un futuro, anche economicamente sostenibile, a questo Paese. I giovani di oggi non hanno bisogno di votare anche per il Senato; i giovani di oggi, cari colleghi, hanno bisogno di trovare posti di lavoro. E i posti di lavoro si trovano se la macchina funziona, se le istituzioni funzionano, se l'economia cresce, se l'occupazione cresce in conseguenza della crescita della nostra economia e delle nostre imprese. Stiamo marciando male. Questa storia, che domani avrà due righe sui giornali, caro collega Castaldi, dopodomani già l'hanno dimenticata tutti, a cominciare da quei diciottenni che forse neanche andranno a votare. *(Applausi)*. Sì, è vero, Sì, è vero, ci sono circa quattro milioni di italiani collocati fra l'elettorato attivo alla Camera e l'elettorato passivo al Senato, secondo i dati del servizio Studi del Senato della Repubblica ricavati dalle ultime elezioni del 2018. Benissimo, ma c'era una ragione per la quale i nostri Padri costituenti hanno ritenuto che la Camera e il Senato avessero ruoli differenti, per cui l'elettorato attivo e l'elettorato passivo dovessero essere diversi. Certamente sì, non erano mica dei sottosviluppati. Tanto è vero che, guarda caso, in tutte le Commissioni bicamerali, da quella Bozzi a quella D'Alema e via di seguito, l'unica che ha comunque previsto un adeguamento era quella che prevedeva un ridisegno del nostro ordinamento costituzionale, con una nuova logica nella quale Camera e Senato dovessero fare cose differenti perché vi sarebbe stato il superamento del cosiddetto bicameralismo paritario. Tutto questo però oggi non c'è c'è perché non si riforma la Costituzione in questo modo. È sbagliato e lo dico da umile servitore e studioso della nostra Costituzione.

Mi sono spiegato? Alla fine chi interverrà in dichiarazione di voto, forse dirà che ci asteniamo; io sono contro i voti di astensione, però mi adeguo. Permettetemi di dire che io avrei votato sinceramente contro il provvedimento perché per me è sbagliato.

da quando è nato questo Governo di unità nazionale, esiste la speranza di un futuro che possa superare il populismo e la demagogia, la ricerca del consenso andando a grattare i mal di pancia dei cittadini e delle cittadine. Mi auguro che tutto questo venga superato e che per l'Italia possa esserci un futuro migliore rispetto a riformette da quattro soldi come quella di

Presidente, colleghi, siamo chiamati a votare una riforma costituzionale epocale. Dopo settantacinque anni dalla nascita della Repubblica e del riconoscimento del diritto di voto a tutti i cittadini, donne comprese, finalmente lo stesso diritto ad un voto libero, personale, uguale e segreto, viene riconosciuto a 4,5 milioni di giovani di età compresa tra i diciotto e i i quali potranno votare i senatori della Repubblica. Si tratta dunque di una riforma che riconosce pari dignità a tutti i cittadini, maggiorenni compresi, ad esercitare i loro diritti politici e quindi a partecipare attivamente alla vita politica del Paese. Dopo una lunga recessione economica che ha visto i giovani tra i soggetti più vulnerabili e la pandemia che li ha costretti ad ulteriori restrizioni dei loro diritti costituzionali, come il diritto allo studio, ai movimenti, alle attività e alle relazioni sociali, siamo davvero orgogliosi come parlamentari di approvare oggi una riforma che aspettavano da tempo, la quale restituirà loro maggiore fiducia nelle Istituzioni e ridurrà l'astensionismo nelle competizioni elettorali. I giovani hanno voglia di tornare alla vita e di dare un contributo concreto alla vita politica e sociale del Paese. nostro esame che riduce l'età dell'elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica si inserisce in un più ampio percorso di riforme costituzionali, iniziato con il taglio di un terzo dei parlamentari, portato a casa da questa legislatura. L'obiettivo è rendere il Parlamento un'istituzione snella ed efficiente, senza dover rinunciare alla rappresentanza territoriale dei cittadini. Per questo consentire a 4,5 milioni di giovani di scegliere con l'esercizio del diritto di voto i senatori della Repubblica non significa dover rinunciare a una Camera del Parlamento. Il bicameralismo perfetto, e quindi un sistema legislativo fondato su due Camere aventi ciascuna gli stessi poteri, deve restare un nostro pilastro costituzionale perché ciò non significa perdere tempo, come sostiene qualcuno. La doppia lettura di un testo di legge non è un'inutile ripetizione, ma serve a impedire un'approvazione frettolosa di testi di legge che poi devono essere corretti da un altro legislatore oppure, come spesso accade, modificati dalla giurisprudenza. Ciò avviene con un enorme aggravio del lavoro della magistratura che, come abbiamo visto in questi anni, comporta ingenti spese per il sistema giustizia nel peggiore dei casi, denegata giustizia. Questo è il motivo per cui, durante i lavori della riforma costituzionale, si è scelto di non modificare l'età dell'elettorato passivo, lasciando che il Senato resti la Camera alta, la Camera dei saggi e della politica più matura. Ciò non vuole essere un'esclusione di una parte della società civile, ma lo stimolo a impegnarsi nella vita professionale e politica per raggiungere traguardi più impegnativi. concludo con l'auspicio che i nostri giovani siano sempre più coinvolti nella vita politica del Paese e che le loro esigenze siano poste in primo piano, così come è voluto oggi dal PNRR, al fine di garantire loro le dovute attenzioni in tutti i settori della vita civile, dal lavoro, all'istruzione, alla cultura e all'educazione. Con il riconoscimento del diritto di voto al Senato certamente torneranno ad avere una maggiore fiducia nei politici, nella politica e nelle istituzioni. *(Applausi)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, sarò quasi telegrafico perché il collega Pagano ha chiarito in maniera inequivocabile la nostra posizione e, soprattutto, ha chiarito la battaglia che in 1a Commissione io e lui ci siamo trovati a sostenere

Il problema non è modificare la Costituzione, ma farlo rendendo la nostra impalcatura istituzionale coerente, funzionale, efficiente e rapida. Non mi sembra che procedendo di questo passo si abbia un progetto organico che possa poi servire a sveltire, semplificare e rendere efficiente il nostro sistema. sistema. Durante la discussione in Commissione affari costituzionali a proposito della riduzione del numero dei parlamentari, il presidente Calderoli ebbe a dire, di fronte a una critica sul modo di operare in maniera settoriale le riforme costituzionali, che ormai si era convinto

d'accordissimo che è necessario agire in questa maniera, ma in un contesto complessivo nel quale sappiamo dove dobbiamo arrivare. Abbiamo ridotto il numero dei parlamentari senza modificare i Regolamenti parlamentari e senza modificare la legge elettorale. *(Applausi)*. Abbiamo allontanato i cittadini dalla politica, altro che interessare i cittadini e i giovani alla politica! Con questa riforma si fa un altro *slogan*, che non si sa dove ci porta.

che in campagna elettorale era stato avvicinato da moltissimi giovani che gli chiedevano: quando sarà possibile per noi diciottenni votare per il Senato? Personalmente non ne ho incontrato nessuno,

non si tratta di dare legittimazione al mondo giovanile, che con la riforma del 1975 ha già una legittimazione elettorale: elegge la Camera dei deputati.

estendiamo alla stessa platea la possibilità di eleggere la Camera e il Senato, una delle due Camere è assolutamente inutile, non serve a nulla. Volete estendere il voto ai diciottenni? Benissimo, fatelo, ma allora abrogate il Senato o abrogate la Camera, perché questo significa ottimizzare, anche in una prospettiva di *spending review*. Si parla di tagli in questo momento, i vitalizi, chissà quanti risparmi si faranno, e invece sono questi i veri risparmi strutturali che possono servire al Paese. Abbiamo una Camera di troppo, facciamocene una ragione. Allora, vogliamo far votare per il Senato? Benissimo, abroghiamo la Camera dei deputati. Non lo volete fare? Allora il Senato deve avere gli stessi rappresentanti che ha la Camera dei deputati altrimenti queste riforme non sono inutili, sono irrazionali, non si capiscono. Non Non so a quanti di voi è capitato: ogni tanto, la sera faccio *zapping* sui programmi televisivi e ci sono alcune inchieste giornalistiche nelle quali

Veramente qui c'è qualcosa che non funziona, come diceva il collega Pagano. Caro collega, non ha importanza il fatto che siamo stati soccombenti sia nella battaglia per difendere la struttura

non è una maggioranza politica che si è creata intorno a una prospettiva; è una maggioranza occasionale che si trova d'accordo su una riforma, ripeto, non inutile, ma irrazionale. Collega Pagano, non non dobbiamo darci pena del fatto di essere stati soccombenti, perché nella vita non è importante sostenere le battaglie che si vincono; è importante sostenere le battaglie nelle quali si crede. *(Applausi)*. Noi in queste battaglie crediamo e probabilmente, un giorno, qualcuno, leggendo i Resoconti parlamentari, ci potrà dare quella ragione che oggi ci è stata negata. Anche io, cara presidente Bernini, sarei stato più portato a votare contro, ma la differenza è relativa, anche perché non voglio che domani si scriva sui giornali che siamo contro i giovani. Noi siamo a favore dei giovani, le nostre politiche economiche giovanili sono all'avanguardia, nell'interesse di quanto serve ai giovani. Quindi, la nostra astensione è un voto contemporaneamente di protesta verso questo modo di agire e anche un segnale al mondo giovanile, al quale sicuramente vogliamo riconoscere diritti ma anche doveri. Sono stato tra i sostenitori dell'opportunità di reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Mi auguro

non si abbiano volti stravolti o risposte strampalate, bensì risposte adeguate. Quando avremo raggiunto questo grado di cultura, di civismo e di diritto di cittadinanza, forse questa riforma potrà essere idonea; ma in questo momento, secondo il nostro modesto avviso, è assolutamente inutile. Ciò nonostante, ci asterremo su questo provvedimento perché non vogliamo contribuire a violentare ingiustamente la nostra Costituzione.

Signor Presidente, Governo, colleghi, poche settimane fa, in occasione di una discussione che riguardava sempre la modifica della Costituzione, ho sostenuto che serve cautela nell'avviare un *iter* in tal senso. Serve cautela, serve valutare l'opportunità serve valutare le conseguenze dell'atto che si va ad approvare. E questo non perché, come molti qui dentro, ma anche moltissimi al di fuori di questa assise, creda che la nostra sia la Costituzione più bella del mondo. Questo non lo penso assolutamente; io ritengo che in alcune parti la nostra Costituzione sia anacronistica e non potrebbe che essere così. Essa è stata adottata quasi settantacinque anni fa, in un contesto storico-sociale

non può che essere anacronistico ora o essere stato eccessivamente futuristico allora. Questo avrebbe significato che i Padri costituenti abbiano commesso degli errori; ma questo non lo penso assolutamente. Quindi, la nostra Costituzione può e deve essere modificata; lo abbiamo fatto di recente e lo stiamo facendo anche adesso. Ciò non toglie però che essa, seppur appunto anziana (consentitemi il termine), abbia comunque in sé dei principi assolutamente condivisibili. per me, uno dei principi più importanti in assoluto contenuti nella Costituzione, al secondo comma dell'articolo 1, è quello che prevede che la sovranità spetti al popolo, che la esercita nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione. Che significa questo? Significa che il potere (perché parlando di sovranità di questo si tratta) spetta al popolo, che tramite i propri rappresentanti eletti, quindi tramite il voto, esercita questo diritto. Perché ritengo di dover precisare questo aspetto? Innanzitutto perché la discussione odierna verte su uno di questi aspetti, appunto il fatto che l'esercizio del voto sia disciplinato sia con riferimento all'elettorato passivo, sia con riferimento all'elettorato attivo. Per la prima fattispecie è prevista una differenza di età per poter accedere alla Camera dei deputati o essere eletti al Senato; con riferimento invece all'elettorato attivo, sono previsti due livelli di età diversi per poter scegliere i propri rappresentanti eletti. Di nuovo quindi parlo di rappresentanti eletti e non lo faccio a caso, come non a caso ho ricordato a chi la nostra Costituzione attribuisce il potere. Ritengo infatti gravissimo che un organo costituzionale, tramite i propri rappresentanti (in questo caso sto parlando dell'Associazione nazionale magistrati), arrivi a pronunciarsi contro un'iniziativa del primo partito d'Italia, che chiede semplicemente al popolo, cioè a colui che detiene il potere, di esprimersi sull'opportunità di poter coinvolgere tutta la popolazione su un *referendum*. Sostanzialmente un ordine dello Stato si oppone a far sì che chi detiene detiene il potere per previsione costituzionale si possa pronunciare su un tema così importante per il nostro ordinamento giuridico. Questo è gravissimo. Come dicevo prima, un ordine dello Stato, perché molti, anche qui dentro, ritengono, a mio avviso impropriamente e sbagliando, che il potere esecutivo, uno dei tre poteri unanimemente riconosciuti (insieme al legislativo e al giudiziario), sia titolarità della magistratura. Ma così non è. La nostra Costituzione, oltre a dire che il potere spetta al popolo, all'articolo 104 dice chiaramente che la magistratura è un ordine. Quindi, un ordine non dovrebbe consentire la limitazione dell'esercizio del potere a chi legittimamente lo detiene. Ma noi andiamo avanti: andiamo avanti nelle piazze, dove siamo sempre stati e continueremo ad esserci, e andiamo avanti nei gazebo, che abbiamo sempre fatto e continueremo a fare.

non solo tutta la mia solidarietà e vicinanza, ma anche i miei sentiti ringraziamenti a loro e a tutti gli altri militanti che hanno consentito di realizzare più di 1.000 gazebo e di raccogliere più di 100.000 firme a sostegno di questa iniziativa di democrazia. Questo perché la Lega, soprattutto nei momenti di difficoltà, è in mezzo alle persone. Molti, nei momenti di difficoltà, si chiudono nel palazzo, si arroccano; noi, al contrario, scendiamo nelle piazze. Ne sono testimone diretto: quando il precedente Governo ha limitato le attività, ho preso un impegno per cui poco più di un mese fa ero a parlare con il generale alla base (e il generale non è un militare e la base non è una caserma, ma una palestra). Nel momento in cui il precedente Governo limitava

Senato. Dicevo che ritengo utile questa previsione perché, quando è stato adottato questo limite, il contesto storico-sociale era completamente diverso: si era appena raggiunto il suffragio il suffragio universale, quindi la possibilità di far votare anche le donne; pochi anni prima però, fino al 1912, nemmeno tutti gli uomini potevano votare, perché occorreva avere un certo livello culturale ed essere espressione di una certa classe sociale.

anziché ridursi, è addirittura aumentata, perché, quando è stata adottata la Costituzione, la maggiore età si conseguiva a ventun anni, quindi la differenza tra chi poteva votare per la Camera e chi per il Senato era di quattro anni; successivamente, con l'abbassamento della maggiore età a diciotto anni, questa sperequazione è aumentata, tanto che in questo momento la differenza è di sette anni. Una conseguenza diretta è stata che alle ultime elezioni

Allora, se dobbiamo perseguire l'interesse delle future generazioni, è utile, è opportuno ed è bene che queste si facciano partecipi anche delle decisioni. A differenza di alcuni colleghi che credono che questo sarebbe in contraddizione con una situazione di fatto che prevede una certa ignoranza diffusa

quasi in obbligo civile di essere più partecipi all'attività democratica del proprio Paese. Ci sarebbero state ulteriori questioni, ma il tempo sta per finire, quindi concludo il mio intervento ringraziando per l'attenzione ricevuta.

signori membri del Governo, sono oltre quarantacinque anni che si discute in Parlamento dell'opportunità di ridurre i requisiti di età per l'elettorato attivo. Le proposte, nel corso delle diverse decadi, sono pervenute da parte di tutti gli schieramenti dell'arco parlamentare, dal MoVimento 5 Stelle e, ben prima, dal Partito Democratico e anche dalla Lega. Molto è stato detto, sono stati realizzati iniziative, studi e ricerche sull'elettorato giovanile, si sono confrontate diverse proposte che però non sono mai giunte al termine del percorso parlamentare. Oggi si cambia storia: finalmente portiamo a termine una riforma semplice, chiara, in linea con lo stile che abbiamo inaugurato in questa legislatura, quello delle riforme costituzionali puntuali. Penso alle altre proposte presentate dal MoVimento 5 Stelle, che hanno innovato la Costituzione, come la riduzione del numero dei parlamentari, che è stata approvata anche a larga maggioranza dalla popolazione. Come detto, questo disegno di legge è davvero molto semplice: con un solo comma riconosciamo ai giovani tra i diciotto e i venticinque anni il diritto di esprimere il loro voto non solo per la Camera, ma anche per il Senato, come succede nella maggior parte degli Stati europei con bicameralismo. I giovani sono i nostri concittadini, la parte più vitale e propositiva della cittadinanza, che fino ad oggi ha contato a metà, quando si trattava di scegliere i rappresentanti eletti del popolo italiano. Dare loro la possibilità di votare anche per il Senato significa affermare chiaramente un principio democratico basilare e potenziare i diritti politici di ben quattro milioni di persone. La crisi economica, sociale e ambientale che stiamo vivendo è il frutto delle scelte politiche ed economiche che sono state fatte negli scorsi decenni. Allo stesso modo, le scelte politiche di oggi condizioneranno fortemente in positivo o in negativo il nostro futuro e chi ha più a cuore il futuro, se non i giovani? Coloro che più di tutti pagheranno o beneficeranno delle scelte politiche di oggi sono i giovani, che hanno tutta la vita davanti. Ecco perché è giusto che il loro voto sia pari e non dimezzato rispetto a quello dei loro genitori e dei loro nonni. È giusto che possano incidere pienamente sul futuro del Paese. Non solo, dare voce ai giovani significa dare loro fiducia, importanza e responsabilità. Sono convinta che sia un passo importante per spronarli a partecipare sempre più consapevolmente alla vita politica del Paese. Inoltre, con il voto dei giovani per il Senato si compenserà, almeno in parte, l'enorme peso elettorale della popolazione più anziana.

Peraltro, il *quorum* di elettorato attivo diverso tra Camera e Senato è stato una delle cause della costituzione di maggioranze diverse tra i due rami del Parlamento, che spesso nella nostra storia ha condotto all'ingovernabilità. Questa riforma risolve, quindi, uno dei problemi e garantisce una migliore stabilità di tale istituzione. In conclusione, colleghe e colleghi, oggi un diciottenne può lavorare, guidare una macchina, contrarre matrimonio, comprare una casa, stipulare contratti e aprire un conto in banca, quindi non si capisce perché mai non possa esprimere un voto pieno per il Parlamento, scegliendo i propri rappresentanti in Senato. Ai giovani dev'essere data fiducia. Innanzitutto, l'educazione deve restituire loro la fiducia in se stessi. Purtroppo, oggi l'educazione impartita ai giovani sminuisce e svilisce la loro autostima, mentre, al contrario, essa deve trasmettere fiducia, sicurezza e anche la consapevolezza che si devono prendere decisioni assunzioni di responsabilità e che, se malauguratamente si sbaglia, c'è la possibilità di riconoscere i propri errori e di correggerli. Abbiamo quindi un grande bisogno dei giovani. La loro freschezza, la loro energia, la loro sensibilità e la loro consapevolezza dei problemi globali che dobbiamo affrontare sono qualità preziose, soprattutto in un momento storico che chiede grandi cambiamenti in tempi brevissimi. L'inclusione dei diciottenni nell'elettorato attivo per il Senato preannuncia questa apertura alle innovazioni e ai cambiamenti che sono in corso nel nostro secolo.

promossa da Coldiretti sul tema della mobilitazione della fauna selvatica, a cui partecipano il ministro Patuanelli,

sono poi anche Presidenti di Regioni, come Michele Emiliano, Governatore della Regione Puglia, Stefano Bonaccini, Governatore della Regione Emilia-Romagna, e altri. C'è anche l'assessore all'agricoltura della Regione Campania. Ci saranno quindi esponenti di tutte le parti politiche. Sarebbe interessante che si desse un segnale di attenzione al tema, inserendo nel calendario una risoluzione, che tra l'altro è stata approvata a larga maggioranza, con la sola astensione - lo dico in termini corretti - dei cinque esponenti del MoVimento 5 Stelle, in Commissione agricoltura.

causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica. La discussione in Assemblea, tra l'altro, è stata anche richiesta dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento. Ne avevo accennato ieri in sede di Conferenza dei Capigruppo.

su cui mi dissocio dalla proposta del senatore Romeo, è che non possiamo presentare un'altra risoluzione, purtroppo, e quindi abbiamo la necessità di di preparare un ordine del giorno per affiancarlo alla discussione, che potrà essere votato dopo la risoluzione stessa. Per questo motivo, avanziamo una richiesta un po' complicata, visto che domani facciamo le riforme costituzionali:

portatori di interessi, gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori, perché questo è un problema che un falso ambientalismo e un falso animalismo hanno sempre tentato di mettere Oggi abbiamo la possibilità, con questa risoluzione, approvata - come diceva il capogruppo Romeo - in Commissione agricoltura senza alcun voto contrario, alla fine di un percorso lungo e intenso, di dare una risposta agli agricoltori e agli allevatori su un problema che ormai è diventato

Signor Presidente, non voglio ripetere cose già dette in maniera egregia dai colleghi, ma non ritengo si tratti di una forzatura, visto che di questo si è parlato tanto anche nei giorni scorsi, perché da tempo il tema è all'ordine del giorno e dei lavori della Commissione agricoltura e, come hanno ricordato i colleghi, la risoluzione è amplissimamente condivisa, nei termini di maggioranza qualificata richiesti per farla arrivare immediatamente in Aula. Altro non siamo quindi, in questo momento, che interpreti di una volontà espressa dalla Commissione, con la maggioranza qualificata richiesta, che coincide con un momento importante per l'agricoltura

Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle per aderire a quanto dichiarato dalla collega De Petris in ordine alla nostra volontà di elaborare un ordine del giorno alternativo. Pertanto, chiediamo qualche giorno per arrivare a un testo che abbia senso compiuto. Da componente della Commissione agricoltura, mi permetto di dire che quello svolto dal collega La Pietra è stato un lavoro lungo e meticoloso, con il tentativo di includere le volontà che erano espressione della Commissione. Cionondimeno, non si è addivenuti ad un testo condiviso e ricordiamo che il Governo ha posto un'ipoteca su quel testo esprimendo un parere negativo del quale non abbiamo potuto non tenere conto, tant'è che ci siamo anche astenuti in Commissione per non arrivare a una rottura completa. Ciò detto, ripeto che chiediamo ancora qualche giorno per elaborare un ordine del giorno alternativo.

l'egregio lavoro che abbiamo fatto in Commissione agricoltura (ma non è una novità e ce lo siamo detti più volte in quest'Aula: abbiamo la capacità di lavorare bene, di approfondire i temi

prendere un po' di tempo *(Commenti)*, come hanno chiesto sia la presidente De Petris sia il collega Trentacoste del MoVimento 5 Stelle, cercando di trovare ancora una volta su questo tema importante per i nostri

**Il Senato non approva**.